L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Onorevoli colleghi, il gravissimo terremoto che ha colpito, nella notte tra domenica e lunedì, la città dell'Aquila ed i suoi dintorni ha suscitato nel Paese e nel mondo un moto di cordoglio e di profonda commozione. Tutta l'Italia ha chinato il capo di fronte all'atroce numero di vite spezzate dalla violenza del sisma, ed ha trepidato per la sorte delle tante persone rimaste intrappolate tra le macerie. Al dolore per le vittime, tra le quali si contano purtroppo anche tanti bambini, ed alla speranza di salvare ancora quante più vite è possibile, alimentata dalla prontezza con la quale si è sin dalle prime ore dispiegata la macchina dei soccorsi, si è affiancato un sentimento di viva preoccupazione per i destini di migliaia di famiglie che, in quella terribile notte, hanno perduto i beni e i riferimenti più importanti della loro vita personale e collettiva. Centinaia di persone sono state duramente colpite nella salute e negli affetti più cari e migliaia di nostri concittadini hanno visto svanire nella polvere la loro casa, il loro posto di lavoro, tutti quei luoghi e quegli edifici che costituiscono il simbolo e l'anima di ogni comunità: la scuola, la chiesa, il municipio, l'ospedale. Nei giorni scorsi avevo pensato subito di recarmi in Abruzzo, per portare la solidarietà del Senato della Repubblica alle popolazioni così duramente colpite da questa immane tragedia, ma ho poi preferito rinviare, per non recare intralcio al difficile lavoro dei soccorritori in questa prima, delicata fase degli interventi e delle ricerche dei dispersi. Mi recherò quindi, in uno dei prossimi giorni, nelle zone del sisma per manifestare la vicinanza di noi tutti ai nostri fratelli abruzzesi. I Capigruppo hanno poco fa convenuto con la proposta da me avanzata di prevedere un contributo di almeno 1.000 euro a senatore, più eventuali somme aggiuntive che il Gruppo vorrà mettere a disposizione, da destinare ai bambini vittime di questa tragedia. A tale riguardo è con piacere che comunico all'Assemblea che i colleghi senatori a vita Carlo Azeglio Ciampi ed Emilio Colombo mi hanno informato di voler destinare i propri emolumenti parlamentari del mese di aprile alla sottoscrizione. Analoga sottoscrizione sarà organizzata dall'Amministrazione del Senato. Per superare questa durissima prova, il popolo abruzzese potrà quindi contare, oltre che sulle sue antiche doti di coraggio e di tenacia, sul sostegno assiduo e compatto dell'intera comunità nazionale. Questo accadrà non soltanto nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, come ha dimostrato l'ondata di solidarietà che si è sviluppata in tutte le Regioni d'Italia, con i cittadini pronti a mettersi in fila per donare il sangue o per offrire agli sfollati un riparo temporaneo nelle proprie case. Ma dovrà accadere anche nella fase successiva, meno coinvolgente sul piano emotivo ma altrettanto urgente e drammatica, che porrà le istituzioni nazionali, regionali e locali di fronte al difficile compito di ricostruire le case e i centri squassati dalla forza del terremoto, di far ripartire le attività economiche e di recuperare al meglio quel tessuto urbanistico e civile e quegli straordinari tesori d'arte e di storia che oggi si rivelano gravemente danneggiati, se non completamente distrutti. Lo si potrà fare se si saprà fare tesoro dell'esperienza del passato, valorizzando il ruolo determinante delle autonomie locali nella ricostruzione, in un quadro di piena e vera solidarietà nazionale per le necessità primarie di territori così duramente colpiti dalla natura. Sono certo che su questi temi fondamentali si conserverà l'unità tra tutte le forze politiche, che con grande responsabilità si sono strette, in queste ore, intorno alle istituzioni che stanno concretamente operando, manifestando la volontà di mettere le proprie energie e le proprie strutture a disposizione dello sforzo nazionale e di contribuire a sostenere l'azione dello Stato e del Governo. Esprimo, quindi, il sentimento unanime di tutta l'Assemblea nel manifestare un profondo ringraziamento all'azione instancabile delle migliaia di soccorritori che, provenienti da tutte le regioni d'Italia, si dedicano ancora oggi, senza sosta, a ricercare i dispersi, curare i feriti, sgomberare le macerie, rendere sicure le strade, fornire assistenza alle migliaia di sfollati. Rivolgo pertanto un sincero ringraziamento alla Protezione civile, alle forze dell'ordine, ai nostri militari, agli operatori della Croce rossa, agli uomini e alle donne del Servizio sanitario, nonché alle migliaia di volontari che in questi giorni si prodigano per limitare gli effetti della sciagura e lenire le sofferenze delle vittime. Per esprimere la nostra partecipazione al dolore ed al cordoglio dell'intero Paese, sospendo la seduta per dieci minuti in segno di lutto.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento renderà ora un'informativa al Senato sul terremoto in Abruzzo. I rappresentanti dei Gruppi potranno poi intervenire per dieci minuti ciascuno. Si passerà quindi allo svolgimento delle relazioni sul disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure a sostegno dei settori industriali in crisi, già approvato dalla Camera dei deputati. Su tale provvedimento il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha preannunciato l'intento del Governo di porre la questione di fiducia, in relazione all'imminente scadenza. I Capigruppo hanno pertanto già provveduto a organizzare i tempi del dibattito. Per la discussione generale sulla fiducia, che si concluderà entro questa sera, anche oltre l'orario di chiusura già previsto, sono state ripartite tra i Gruppi sei ore. Le dichiarazioni di voto finale si svolgeranno domani mattina con inizio alle ore 9. Pertanto la chiama per il voto di fiducia inizierà intorno alle ore 10. La votazione per l'elezione di due componenti del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, già prevista per oggi alle ore 12, è stata rinviata alla ripresa dei lavori dopo le festività pasquali. Resta confermato che nella settimana dopo Pasqua l'Assemblea non terrà seduta. Peraltro, nel corso di tale settimana potranno convocarsi le Commissioni in relazione ai rispettivi programmi dei lavori, con particolare riguardo agli argomenti iscritti nel calendario dell'Assemblea, nonché ad attività connesse ad interventi relativi al terremoto in Abruzzo. L'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 21 aprile per la discussione del decreto-legge in materia di atti persecutori, attualmente all'esame della Camera dei deputati. Nel corso di tale settimana saranno inoltre poste all'ordine del giorno mozioni sugli italiani nel mondo, sulle mine antipersona, sui trasporti ferroviari nel Mezzogiorno e sull'embargo a Cuba. Mercoledì 22 aprile alle ore 12 si procederà alle votazioni per 1'elezione di due componenti ciascuno nei Consigli di presidenza della Giustizia tributaria, della Giustizia amministrativa e della Corte dei conti. Giovedì 23 aprile si voterà per 1'elezione dei quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti. Nella settimana successiva, a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 28 aprile, sarà discusso il disegno di legge collegato sul federalismo fiscale. Successivamente si passerà all'esame del disegno di legge collegato su internazionalizzazione imprese ed energia. Nella seduta pomeridiana di giovedì 30 aprile si svolgeranno interrogazioni a risposta immediata su materie che saranno segnalate dai Gruppi.

Signor Presidente, come è noto nella notte tra il 5 e il 6 aprile, alle ore 3,32, un fenomeno sismico di magnitudo 5,8 grazie In particolare, nella giornata di ieri 7 aprile e nella scorsa notte si sono verificate ulteriori scosse, di cui le più rilevanti si sono manifestate rispettivamente alle ore 11,38 (di magnitudo 4,7), alle ore 19,47 (di magnitudo 5,3) e alle ore 23,34 (di magnitudo 4.2). L'evento sismico ha purtroppo provocato crolli diffusi in numerosi Comuni della Provincia dell'Aquila ed in altri Comuni della Regione Abruzzo, causando la perdita di numerose vite umane, numerosi feriti e, data l'estensione dell'evento, il conseguente sgombero di numerosissimi immobili. Ad oggi, il numero dei decessi è purtroppo salito a 250, di cui nel pomeriggio di ieri 17 vittime risultavano ancora in attesa di identificazione da parte della polizia scientifica e dal GIS dell'Arma dei carabinieri. Data la gravità della situazione, per interpretare il sentimento diffuso in tutto il Paese di profonda commozione, il Consiglio dei ministri si accinge a dichiarare per le prossime giornate una giornata di lutto nazionale. Attualmente i dispersi risultano 11, i feriti allo stato 1.179, di cui 179 più gravi e perciò trasferiti in strutture ospedaliere fuori della Regione. Circa 150 infine - questa è la notizia più sollevante - sono state le persone estratte vive dalle macerie. La notizia della gravità dell'evento ha superato i confini nazionali tanto che sinora sono state 35 le Nazioni che hanno offerto al nostro Paese la propria solidarietà nel fronteggiare un'emergenza così grave. Darò ora conto, Presidente, dello straordinario impegno e dell'immediata attivazione da parte del nostro sistema della Protezione civile e dello straordinario impegno che si sta ininterrottamente manifestando dalle ore 4 dell'altra notte da parte di tutti gli uomini delle Forze armate, delle forze dell'ordine, Polizia e Carabinieri, Guardia di finanza, Corpo forestale, Vigili del fuoco e degli uomini del volontariato. A queste straordinarie persone, Presidente, a nome del Governo, ma so di poter interpretare anche il sentimento suo, dell'Assemblea e del Paese, intendiamo rivolgere il nostro più sentito ringraziamento. A seguito dell'immediata comunicazione da parte dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia relativo all'evento sismico sono state immediatamente contattate tutte le sale operative delle strutture presenti nella sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile e, data l'estrema gravità della situazione apparsa subito tale, alle ore 4 del 6 aprile è stato convocato il Comitato operativo della Protezione civile, presieduto dal dottor Guido Bertolaso, a cui hanno partecipato tutti i rappresentanti delle componenti e delle strutture operative di Protezione civile. Da tale momento la riunione del Comitato operativo è stata ininterrottamente attiva, e lo è tuttora. Dalle prime ed immediate verifiche effettuate sul territorio sono stati registrati crolli in particolare nel centro storico del capoluogo aquilano ed in numerosi centri minori e limitrofi all'Aquila, tra i quali maggiormente a Paganica, Fossa e Poggio Licenze. Successivamente si è avuta notizia della quasi totale distruzione del centro storico di Onna**.** Nel corso della mattina sono subito partiti nove nuclei di Protezione civile diretti nelle località maggiormente colpite e sono state attivate tutte le colonne mobili dei Vigili del fuoco - che intendo qui ringraziare - da tutte le Regioni italiane, ad eccezione naturalmente di quelle della Sicilia e della Sardegna per evidenti ragioni logistiche. Presso la sede della scuola della Guardia di finanza dell'Aquila è stata istituita la Direzione comando e controllo e successivamente all'Aquila, San Demetrio, Pizzoli, Rocca di Mezzo e Paganica sono stati istituiti 5 centri operativi misti che ospitano 31 aree di ricovero.

Alle ore 7,30 il dottor Bertolaso, accompagnato dal vice capo della Polizia, dal commissario della Croce rossa italiana, dal capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da un ulteriore *team* del Dipartimento nazionale della protezione civile, ha effettuato la prima ricognizione in elicottero sulle aeree interessate dal sisma, mentre sono stati attivati i primi interventi di assistenza alla popolazione colpita. Sono state allestite 20 tendopoli per un totale di più di 2.416 tende per ospitare fino a 14.500 persone. Si è provveduto ad assicurare la distribuzione giornaliera di circa 18.000 pasti, assicurati da 25 cucine da campo e le persone attualmente assistite sono circa 18.000. Inoltre, già dal 6 aprile la città di Pescasseroli ha reso disponibili 4.000 posti letto in alberghi e campeggi per gli abitanti della Provincia dell'Aquila ed al momento risulta che 907 persone sono ospitate in strutture alberghiere. Per quanto riguarda le risorse messe a disposizione dalle strutture operative di protezione civile impegnate in emergenza, si evidenzia che al 7 aprile il numero del personale del Dipartimento della protezione civile impiegato nell'attività di coordinamento e verifica dei danni risultava essere di circa 110 unità, mentre il numero delle forze impiegate dall'intero sistema di Protezione civile ammonta a circa 8.000 con la presenza di persone provenienti da 12 Regioni. Dalle prime ore del mattino del 6 aprile erano disponibili al decollo 59 mezzi aerei a cui si sono aggiunti 9 mezzi aerei già operativi, diventati rispettivamente il giorno seguente 25 ed 11 sono stati quelli impiegati nell'emergenza. Particolarmente importante è stato l'apporto fornito dalle Forze armate. Tale contributo si è materializzato, sin dalle prime ore dell'emergenza, stante la presenza nella Regione Abruzzo di reparti delle Forze armate dislocati in forma stanziale, con l'intervento di squadre e mezzi specialistici per la ricognizione ed il primo soccorso tratti dal 9° Reggimento alpini e dal 33° Reggimento di artiglieria terrestre "Acqui" con sede all'Aquila e del 123° Reggimento con sede a Chieti. A questi, nel prosieguo dell'emergenza, si sono aggiunti via via assetti specialistici terrestri ed aerei che hanno consentito la costituzione di ben tre *task force* di Esercito, Marina ed Aeronautica, per un totale di 1.530 unità di personale impiegate dotate di 96 mezzi speciali (escavatori, ruspe, torri di illuminazione); 104 mezzi ruotati; 20 elicotteri e 7 aerei (mezzi tuttora impiegati nelle zone colpite dal sisma) Inoltre, l'Esercito, per eventuali ulteriori concorsi in campo sanitario da schierare in zona, ha approntato e resi disponibili un centro sanitario campale per il ricovero e cura ed un posto di medicazione avanzato. Ai suddetti concorsi si è aggiunto l'immediato intervento del personale dell'Arma dei carabinieri, inquadrato nel Comando regionale "Abruzzo", che è stato via via rinforzato da altri 300 Carabinieri provenienti da Regioni limitrofe, nonché dagli assetti specialistici fatti affluire in zona, comprendenti, tra gli altri, 7 unità cinofile per la ricerca di dispersi; 1 nucleo per l'identificazione delle vittime di disastri; un'aliquota del Comando carabinieri per la tutela della salute (in particolare addetta al controllo della salubrità delle acque); 16 stazioni mobili in sostituzione delle caserme particolarmente danneggiate, che sono state dislocate nelle località specificatamente colpite dal sisma; 2 elicotteri impiegati in volo con compiti di ricognizione e trasmissione delle immagini; inoltre, nuclei di collegamento dotati di apparati satellitari avanzati sono anche essi presenti nelle zone colpite dal sisma. è stato particolarmente importante inoltre, sin dall'inizio della gestione dell'emergenza, il ruolo dei Vigili del fuoco. Alle ore 7 del 6 aprile erano già presenti sul posto circa 300 uomini, con circa 100 mezzi operativi. Per effettuare le ricognizioni delle aree sinistrate e per soccorrere i superstiti, alle prime luci dell'alba, appena è stato possibile, sono decollati 4 elicotteri provenienti dai reparti volo di Pescara, Bologna e Roma, con equipaggio integrato con aerosoccorritori dei Vigili del fuoco, specializzati in tecniche speleo-alpinistiche. Nelle ore successive, le forze in campo sono ulteriormente aumentate, sino ad arrivare, intorno alle ore 18, a circa 1.200 unità operative, con oltre 600 mezzi impegnati sul territorio. Contemporaneamente sono state impiegate le colonne mobili operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della Toscana e dell'Emilia-Romagna. Sempre alle ore 18 il Corpo aveva anche reso operativi circa 50 funzionari tecnici specializzati in verifiche della stabilità delle strutture, 40 mezzi speciali movimento terra, 40 unità cinofile, 13 squadre, per un totale di oltre 90 unità specializzate in tecniche speleo-alpino-fluviali, 6 squadre specialistiche per la ricerca delle persone sotto le macerie con attrezzature specifiche di alta tecnologia, quali geofoni, termocamere, attrezzature per il taglio del cemento armato. Moltissime sono state quindi le persone soccorse e messe in sicurezza, delle quali, come dicevo prima, oltre 100 estratte vive dalle macerie. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha allestito quattro campi base presso la scuola della Guardia di finanza, in località Coppito, in provincia dell'Aquila, a Pizzoli-Arischia, nel campo sportivo di Barisciano ed a Monticchio. Alle 18 del 7 aprile, cioè alla data di ieri, risultavano operanti sul territorio colpito dal terremoto 168 sezioni operative provenienti da tutte le Regioni d'Italia, per un totale di 2.386 unità operative, con 83 funzionari tecnici direttivi (ingegneri ed architetti), 13 squadre (per un totale di 90 unità specializzate), 6 squadre specialistiche per la ricerca delle persone sotto le macerie. Vengono attualmente impiegati circa 1.000 mezzi, tra cui 51 mezzi speciali movimento terra e relative strutture di supporto, 24 autoscale, 8 autogru, 30 torri faro, 3 mezzi mobili attrezzati per la trasmissione satellitare, 3 ponti radio mobili e 4 elicotteri. Si sta predisponendo l'invio di 3 autobotti per la fornitura di 52.000 litri di acqua potabile provenienti dai comandi della Campania, 1 autobotte di gasolio per automezzi dal comando di Asti, e 2 autobotti per combustibile avio dai comandi di Bologna e di Pescara. Per quanto riguarda l'impiego delle Forze di polizia, altra struttura operativa, alle ore 14 del 7 aprile scorso nelle zone colpite dall'evento calamitoso, erano presenti 1.724 unità, di cui 566 della Polizia di Stato, 460 dell'Arma dei carabinieri, 318 della Guardia di finanza. Alla stessa data erano anche operative 380 unità del Corpo forestale dello Stato. Per garantire l'ordine pubblico e per le esigenze di soccorso risultano anche impiegate 220 unità dei reparti mobili di Roma, Napoli, Bologna, Bari e della scuola di Senigallia. Sono state impiegate oltre 30 pattuglie per gli interventi di soccorso e la gestione della viabilità, mentre è stato disposto l'invio di ulteriori 26 pattuglie di rinforzo provenienti dai compartimenti del Lazio, delle Marche, della Toscana, della Campania, del Molise e dell'Umbria.

Relativamente, poi, al contributo fornito dal mondo del volontariato, dai dati in possesso del Dipartimento della protezione civile, risulta che nella giornata di ieri il numero delle organizzazioni nazionali di volontariato di protezione per un totale di 941 unità operative presenti *in loco*, raggiunte da un primo scaglione di 245 unità e, successivamente, da un altro scaglione composto da 243 unità, affiancate dalla Croce rossa italiana e dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. A tali forze vanno aggiunti i volontari delle colonne mobili di soccorso aggregati a quelle dei vigili urbani provenienti dalle diverse Regioni del nostro Paese. Il Comune di Roma ha messo a disposizione i mezzi della propria colonna mobile. Per quanto riguarda i servizi essenziali alla popolazione, sulla rete elettrica dell'Aquila già da ieri risultavano disalimentate solo circa 4.000 utenze, mentre si segnalavano criticità limitate relative alla capacità telefonica della rete mobile che si sta provvedendo a ripristinare con interventi di riparazione e di potenziamento finalizzati ad aumentare sensibilmente la capacità di traffico telefonico. La società ENEL ha messo a disposizione 30 gruppi elettrogeni per alimentare una tendopoli da 10.000 persone. Sono stati, inoltre, predisposti mezzi mobili sostitutivi dei servizi postali pronti ad essere inviati *in loco* laddove risultasse necessario, in quanto 51 uffici postali presenti nella zona dell'evento sono in fase di verifica di agibilità post-sisma. L'evento in questione - come sempre accade in questi casi - ha determinato carenze idriche in tutti i Comuni del teramano a nord del comprensorio gestito dall'Azienda acquedottistica, mentre per evidenti ragioni di sicurezza e prudenza la rete del gas è stata disalimentata su richiesta dei Vigili del fuoco. Per quanto concerne la viabilità sulla cui funzionalità, già dal pomeriggio del 6 aprile sono stati avviati gli accertamenti di sicurezza. di sicurezza. Ad oggi la A24 nel tratto Roma-L'Aquila è interdetta solo ai mezzi superiori alle 7,5 tonnellate per facilitare il transito dei mezzi di soccorso, mentre è completamente chiuso al traffico solo il tratto tra Aquila Ovest e Assergi in entrambe le direzioni solo per motivi tecnici. La A25 è ancora interdetta solo al traffico pesante e nel tratto tra Pratola e Bussi Popoli è interrotta per verifiche tecniche. Gravi lesioni strutturali continuano ad interessare la strada statale 5 Tiburtina Valeria, che dal pomeriggio del 6 aprile risulta interrotta dal chilometro 160 al chilometro 169 per la caduta di massi con conseguente deviazione del traffico sulla strada provinciale 9, mentre dal chilometro 176 al chilometro 176,4 è inibita al traffico a causa di un cedimento strutturale in località Corfinio con conseguente deviazione del traffico sulla strada statale 5-dir. Il traffico sulla strada statale 696 risulta tuttora rallentato per la presenza di massi sulla carreggiata e la strada statale 81 in località Penne S. Andrea per la presenza di una chiesa pericolante. Per quanto concerne il traffico su rotaia, lo stesso pomeriggio le Ferrovie dello Stato hanno comunicato che rimaneva interrotto il traffico sulla linea proveniente da Sulmona e su quella per L'Aquila,

a seguito di quella manifestatasi alle ore 23,34, le Ferrovie dello Stato hanno dovuto provvedere a verificare lo stato di sicurezza di alcuni ponti della Provincia, bloccando il transito di quattro convogli di cui uno prima del ponte ferroviario che insiste sul tratto di territorio sito tra Scafa e Torre dei Passeri. In proposito, preme evidenziare che la società della rete Ferrovie italiane ha messo a disposizione otto carrozze letto e una carrozza ferroviaria per la preparazione di pasti caldi, nonché due treni, situati rispettivamente uno a Pescara e l'altro a Roma, con la possibilità di ospitare circa 400 passeggeri ciascuno. partire dalla giornata odierna verrà avviata l'attività di analisi, verifica e stima dei danni. Per effettuare, dunque, la verifica dell'agibilità degli edifici è stata costituita una commissione mista che, per le relative operazioni potrà contare sulla collaborazione di 1.000-1.500 tecnici specializzati, composta anche da rappresentanti del Ministero dei beni culturali per i danni che sono stati recati allo straordinario patrimonio artistico, archeologico e culturale della nostra Regione Abruzzo. Queste sono state le immediate iniziative, tuttora in corso, assunte sul fronte del soccorso e della verifica dei danni. Darò ora brevemente conto, Presidente e onorevoli senatori, delle iniziative assunte dal Governo. Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che ha rinunciato ad andare al previsto *summit* a Mosca per potersi recare già nelle primissime ore del giorno del sisma nel Comune dell'Aquila, per salvaguardare l'incolumità dei cittadini coinvolti e favorire il repentino ritorno alle loro normali condizioni di vita, ha provveduto a nominare nella stessa notte in cui si è verificato il sisma, in qualità di commissario delegato per l'adozione di ogni indispensabile iniziativa, il capo del Dipartimento della protezione civile. Nella stessa giornata di lunedì è stato convocato in seduta straordinaria, e si è riunito alle ore 19, il Consiglio dei ministri, che ha proceduto alla dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992. Il Consiglio dei ministri ha anche provveduto a nominare il nuovo prefetto dell'Aquila, sulla persona del dottor Franco Gabrielli, che ha immediatamente raggiunto la città abruzzese.

Al commissario delegato, dottor Guido Bertolaso, è stato assegnato il compito di assicurare ogni forma di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate, nonché ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale per la salvaguardia delle vite umane. il provvedimento citato autorizza il Presidente della Regione Abruzzo ed i sindaci dei Comuni interessati ad avviare tutte le attività urgenti a garantire il necessario sostegno alla popolazione ed un'adeguata sistemazione per tutti quei cittadini impossibilitati a rientrare nelle loro abitazioni. Presso ciascun Comune sono stati già costituiti gruppi di rilevamento per censire lo stato di agibilità degli edifici pubblici e privati. Tali gruppi sono composti da tecnici qualificati appartenenti alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici. Tra le altre iniziative indispensabili per favorire un rapido ritorno alla vita ordinaria, nell'ordinanza è stata concessa al Dipartimento della protezione civile l'autorizzazione a ricevere e impiegare per i predetti fini

permetta di ringraziare a nome del Governo lei e tutti gli onorevoli senatori per la nobile iniziativa, che ha poc'anzi annunciato, di contribuire in maniera così rilevante a favore delle popolazioni interessate dal sisma.

con straordinarie virtù morali e civili. La prova di coesione e partecipazione civile e morale che sta emergendo deve necessariamente trovare corrispondenza nella risposta che le istituzioni saranno in grado di porre in essere. Ringrazio per questo tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, dell'intero Parlamento per il clima di profondo rispetto, partecipazione e leale collaborazione con il Governo che si sta realizzando in questi giorni.

Signor Presidente, ringrazio il Governo, attraverso il ministro Vito, per le informazioni che ci ha fornito questa mattina e per l'attività svolta in questi giorni. Mi associo a tutte le parole di cordoglio e ai ringraziamenti che lei, signor Presidente, ha formulato in apertura di seduta. La tragedia che si sta consumando all'Aquila e in decine di Paesi del circondario è enorme: le televisioni, la stampa e la rete ci hanno fornito ogni sorta di immagini e racconti strazianti, che non voglio qui commentare, perché a tutti è chiara l'enormità dei danni e delle sofferenze. Oltre ai morti, ai feriti e agli sfollati, voglio richiamare quattro immagini, che a mio avviso simboleggiano più di altre la drammaticità di quanto è accaduto: il crollo del Palazzo del Governo, la Prefettura, che era stata individuata quale sede del coordinamento degli interventi di Protezione civile; la sorte di un grande ospedale, inaugurato meno di dieci anni fa, che doveva essere sicuro per garantire cure immediate alle migliaia di feriti, e che invece è gravemente lesionato e totalmente inagibile; il crollo della Casa dello studente, con la morte di molti ragazzi e di una università dove si stava costruendo il futuro - ora spezzato - di 30.000 giovani e si alimentava una parte importante dell'economia della città; il crollo della Torre medicea di Santo Stefano di Sessanio, uno dei borghi più belli d'Italia, che aveva resistito dal 1200 ad oggi ad ogni sorta di calamità, anche anche sismica, e che rappresentava, più delle altre centinaia di beni culturali distrutti, la possibilità di costruire un futuro per quella economia in grave difficoltà da molti anni. Quattro simboli che connotano l'intensità e la specialità di questa tragedia, che non è solo nel numero dei morti e dei feriti o nell'entità dei danni al patrimonio abitativo e alle infrastrutture, ma nel fatto che, a differenza delle altre simili tragedie, di cui abbiamo viva memoria negli ultimi 40 anni (dal Belice al Friuli, all'Irpinia, fino al Molise, all'Umbria e alle Marche), sono state colpite le funzioni vitali, pubbliche e private, di una città capoluogo di provincia e di regione. Il Comune, la Provincia, la Regione, l'ospedale, l'università e le scuole, gli uffici giudiziari, la prefettura, la questura, i Carabinieri, la Polizia, i Vigili del fuoco, l'ANAS, la Corte dei conti, gli uffici finanziari, l'INPS, l'INAIL e tutti gli altri uffici pubblici sono senza casa e senza mezzi, non possono e non potranno funzionare, non sappiamo per quanto tempo. Il Sindaco, il presidente della Provincia, il questore, il prefetto e quanti altri incaricati di un pubblico ufficio sono senza ufficio e senza casa. Decine di migliaia di attività economiche e professionali hanno totalmente cessato qualunque attività. Anche per questo il terremoto in Abruzzo non è come gli altri e di questo credo non vi sia ancora sufficiente consapevolezza, così come non sono ad oggi calcolabili gli effetti sulla vita anche dei territori non direttamente colpiti dal sisma per effetto della paralisi di molte funzioni pubbliche regionali che avevano sede appunto nel capoluogo di Regione. Nella giornata di ieri, dopo aver visionato con il presidente Marini e con le autorità locali i luoghi del disastro ed aver constatato le atroci sofferenze delle persone, ci siamo a lungo fermati nel centro storico dell'Aquila, una città fantasma, muta e trasfigurata, e ci siamo più volte chiesti quando potrà ripartire. Saranno sufficienti mesi o occorreranno anni? Abbiamo rivolto questa domanda anche al dottor Bertolaso e neanche lui, con la sua esperienza, è stato in grado di fare previsioni. Lo Stato ha risposto prontamente, i soccorsi sono arrivati, anche se ad oggi manca ancora molto: mancano ancora tende e bagni chimici, coperte e molti altri beni. La solidarietà concreta del popolo abruzzese e italiano e di altri Stati, le cui offerte mi guarderei bene dal rifiutare, è stata ed è straordinaria, ma voglio qui oggi annotare che questa volta il programma di rinascita civile ed economica, i progetti di ricostruzione non possono seguire vecchi e lenti riti. Occorrono risorse, soldi veri, probabilmente alcuni miliardi di euro, gran parte dei quali da mettere a disposizione subito o comunque in tempi brevi. Conosciamo le difficoltà del bilancio dello Stato e sappiamo per certo che se non si assumerà questa tragedia come una priorità nazionale, con ogni conseguenza, come ad esempio ritardare altri investimenti infrastrutturali ed altri programmi per poter ottenere l'immediata disponibilità di risorse, non ce la faremo. Prima di parlare di *new town* sarebbe bene pensare e programmare come far ripartire quella città e quella Regione. Noi, il Partito Democratico, abbiamo subito e senza esitazione offerto la nostra collaborazione al Governo ci faremo carico nei prossimi giorni di formulare proposte precise anche di carattere finanziario. Questa disponibilità però non può essere interpretata come remissività. Vigileremo, non ci basteranno le parole, ad ogni impegno dovranno seguire fatti concreti. Ci attende un lavoro duro e noi - statene certi - faremo la nostra parte. Lo dobbiamo a quei bambini e giovani studenti morti; lo dobbiamo all'Abruzzo e a tutto il Paese.

la nostra Regione, il mio Abruzzo. Un ringraziamento particolare e sentito va in primo luogo al presidente Berlusconi e al Governo, il quale ha fatto sentire la sua vicinanza non soltanto con la presenza quotidiana (anche oggi) in Abruzzo, insieme al ministro Zaia, a portare gli della Coldiretti e delle altre organizzazioni ai terremotati, ma anche con un'azione quasi istantanea, se è vero com'è vero che quell'altra splendida figura del Governo, il sottosegretario Bertolaso, dopo poche ore dal sisma è arrivato all'Aquila e ha cominciato un instancabile lavoro di coordinamento e di soccorso che non ha pari e che nobilita l'azione di questo Governo e dell'Italia tutta. Un ringraziamento va alle forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e ai tanti volontari, alle Regioni che ieri, per la prima volta, tutte insieme hanno dato dimostrazione di vicinanza alla nostra Regione. Un ringraziamento particolare, infine, al cuore degli italiani, che si è fatto sentire in tutte le sue forme e in tutti i momenti attraverso la disponibilità a venire in Abruzzo e il desiderio di mobilitarsi.

senza spettacolarizzazioni, seppure nella crudezza del momento, ogni passaggio di queste drammatiche ore, sensibilizzando così l'attenzione dell'Italia, anche oltre i suoi confini. Ci saranno momenti in cui analizzeremo cosa fare. Il Governo ha già annunciato provvedimenti straordinari, a partire dall'immediato aiuto ai processi di ricostruzione, una ricostruzione non soltanto edificatoria ma anche economica, di un'economia che è spezzata, perché questo è un terremoto particolare rispetto a tanti altri che sfortunatamente hanno colpito la nostra Italia. In questo caso, credo per la prima volta, purtroppo, l'epicentro cade in una città capoluogo di Regione, bloccando così non soltanto l'anima ma anche il cuore e il cervello della nostra terra.

approfondire e soffermarci sull'argomento. Io oggi voglio soltanto ricordare qualche passaggio di quanto abbiamo visto, così come diceva poco fa anche il collega Legnini. Tra i tanti drammi che ci sono in queste ore, per chi come me, come lui, come tanti di noi reduci fino a qualche ora fa dalle macerie della città dell'Aquila, credo ci sia un'immagine simbolo di questa tragedia:

questo terribile cataclisma ha spezzato l'esistenza di tanti, ha segnato i percorsi di vita di tutti noi abruzzesi, ha distrutto l'economia di un territorio così vasto, il patrimonio monumentale, quello dei luoghi di culto, la cultura e la storia di una parte dell'Abruzzo. Credo che le immagini di questi giorni abbiano testimoniato che c'è qualcosa che questo sisma non ha potuto spezzare: la dignità e l'orgoglio di un popolo,

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, ringrazio il Governo per l'informativa che ha reso tempestivamente al Parlamento. Vengo anch'io da una Regione che ha vissuto molte volte, troppe, queste tragiche e dolorose esperienze; pertanto il mio primo pensiero va alle oltre 200 vittime e all'immenso dolore dei loro familiari così duramente provati. Permettetemi di esprimere innanzitutto, a nome mio personale e del Gruppo parlamentare che qui rappresento, l'apprezzamento e il sostegno all'azione tempestiva del Governo che sin da subito, sotto il coordinamento della Protezione civile nazionale, ha operato e sta continuando ad operare in modo efficace per la soluzione dei problemi, tanti e drammatici, in cui versa la popolazione colpita dall'evento sismico. L'Aquila per noi diventa la nuova tappa di un lungo calvario che racconta della storia complessa e complessiva del nostro Paese e, permettetemi di dirlo, anche del nostro Mezzogiorno. Dopo Gibellina, Gemona, Sant'Angelo dei Lombardi, Sarno, San Giuliano, dovremo ricordarci di Onna, di Paganica, di Castelnuovo. Vi è quasi un carattere selettivo in queste tragedie ed in questo dolore indicibile che svelano pezzi sconosciuti d'Italia e che raccontano cose su cui dovremmo interrogarci di più quando costruiamo l'agenda della politica. La nostra attenzione non deve però finire nel recinto dell'epicentro e durare lo spazio dell'emozione che rimbalza attraverso il circuito mediatico. Sappiamo che i Comuni coinvolti da questo evento sismico sono molti e che vi è stato un esodo forzato di intere comunità. Il dramma degli sfollati è molto profondo: è il dramma dello sradicamento, soprattutto per i più anziani, che si unisce al dolore indicibile della perdita dei propri cari. L'Italia intera si è stretta intorno all'Abruzzo, ad una comunità che fa del coraggio, della determinazione, dell'orgoglio e della dignità un tratto distintivo del carattere. E all'Aquila in queste ore è stata resa testimonianza di quella trama più intima della nostra coscienza civile che fa giustizia di quegli egoismi che, troppo spesso, sembrano prevalere nel dibattito politico quotidiano. È stato detto che non è questo il momento delle polemiche. È vero. In questi giorni abbiamo potuto vedere concretamente e apprezzare la macchina dei soccorsi, il lavoro instancabile degli operatori della Protezione civile, dei militari delle forze dell'ordine e dei tanti volontari. Abbiamo potuto comprendere anche quanto inutili fossero talune polemiche costruite sui *media*. sui *media*. Polemiche di cartapesta, come quella di dire che questa catastrofe si poteva evitare. Sappiamo bene che non è così. Non lo è mai stato e, forse, non sarà mai possibile evitarlo. Vorremmo però che, spenti i riflettori, non si spegnesse l'attenzione della politica. Non c'è tragedia che non abbia aperto cantieri e avviato una ricostruzione. Nella storia di questo Paese, però, troppe volte il provvisorio è diventato definitivo. E questo non deve più accadere. L'azione del Governo è stata incisiva, sin da subito. Il terremoto, immane tragedia, non deve abbattere insieme alle case le nostre comunità, ma il giorno dopo deve portare con sé una vera occasione di riscatto civile per quelle popolazioni che abitano luoghi a volte ritenuti periferici. Dobbiamo dare il segnale che questo Paese è cresciuto e che la ricostruzione di quel territorio, facendo tesoro dei molti errori del passato, sarà efficace, tempestiva e rispettosa dell'originalità di quei luoghi. Ricordo che dopo un'altra tragedia, quella che sconvolse la comunità di San Giuliano di Puglia, in Molise, l'allora Capo dello Stato, il presidente emerito Ciampi, ebbe a usare parole forti; in particolare disse: «Noi adulti non avevamo provveduto alla sicurezza ed alla protezione dei più piccoli». Vi è da riflettere ancora oggi su tali parole. Tanto più se si pensa che la normativa predisposta subito dopo la tragedia di San Giuliano, a distanza di sei anni da quel terribile evento, non è mai entrata in vigore. Siamo andati avanti di proroga in proroga e ad oggi ancora non l'abbiamo approvata. Questo non è accettabile per un Paese civile e moderno. Ho voluto ricordare le parole del presidente Ciampi perché esse ci aiutano anche a non degenerare nella polemica più più meschina, quella che cerca i ritagli di responsabilità del contingente, quella che vive nello spazio effimero del teatrino di Palazzo. Tuttavia, l'espressione «noi adulti» non è precisa. L'espressione precisa è la seguente: «Le classi dirigenti di questo Paese, ancora una volta, non hanno provveduto alla sicurezza ed alla protezione dei più piccoli». Mi riferisco alla responsabilità di chi pensa che l'opera pubblica di messa in sicurezza del nostro territorio sia soltanto argomento per i dibattiti o per qualche seminario culturale, di chi non riesce a fare una radiografia precisa dello stato delle nostre città, delle nostre coste, delle nostre alture, dei nostri fiumi. Usiamo troppo facilmente l'espressione «calamità naturale». È chiaramente presente un elemento dì fatalità in queste vicende drammatiche, che portano con sé morte e distruzione, tanto più quando si è in presenza di un evento tuttavia, l'espressione «calamità naturale» tante volte è fuorviante, perché la verità è che una parte significativa degli effetti di morte e devastazione derivano da un altro genere di calamità: l'incuria e la disinvoltura umana che quasi sempre è mossa dalla ricerca del profitto personale a danno delle collettività. Attengono alle responsabilità di chi ha vissuto il territorio come un'area di mercificazione o peggio di saccheggio, di chi ha costruito sulle falde e sulla sabbia, di chi ha costruito risparmiando sui materiali di costruzione, di chi ha bucato le alture, di chi ha disboscato, di chi ha inquinato i fiumi. affrontare il dibattito sulla ricostruzione e sul progressivo degrado del nostro Paese, in primo luogo perché ricostruzione significhi, fuori da qualsivoglia manipolazione, rifondazione delle identità ferite, di quel patrimonio prezioso di Comuni piccoli come presepi, che sono lì arroccati nell'Appennino abruzzese e, in secondo luogo, perché il nostro futuro possa essere non sempre e solo governo dell'emergenza, bensì interventi di prevenzione e di risanamento di un territorio così fragile e così esposto a rischi e danni.

Signor Presidente, signor ministro Vito, colleghi senatori, ci uniamo al cordoglio espresso dalla Presidenza nel ricordo delle vittime del violento terremoto che ha colpito l'Abruzzo nella notte tra domenica e lunedì e che procurato danni ingenti alla città dell'Aquila e ai Comuni limitrofi. In questo momento il nostro pensiero e la nostra preoccupazione sono rivolti a quelle tante famiglie colpite dal sisma: a chi ha perso un parente o un amico, a chi ha visto la propria casa ridursi in macerie. A loro esprimiamo solidarietà e vicinanza, oltre a garantire l'impegno nostro e delle istituzioni che rappresentiamo per garantire e assicurare uno standard accettabile di vita in questa situazione di emergenza e per un più rapido possibile ritorno ad una degna quotidianità.

per come hanno lavorato e lavorano in queste ore e questi giorni in Abruzzo, dimostrando un'abnegazione e un attaccamento a valori di solidarietà ed efficienza di gran lunga superiori ai mezzi e alle risorse che si mettono a loro disposizione.

Se il bilancio delle vittime è stato in qualche modo contenuto, se 150 persone sono state estratte vive dalle macerie, l'ultima delle quali a 42 ore dai crolli, lo dobbiamo a loro. Ma un grande contributo sta arrivando anche dalla società civile, dai tanti concittadini che di fronte alle sofferenze dei loro vicini non si sono risparmiati, portando conforto alle persone in difficoltà, aiutando chi è preposto al recupero dei sopravvissuti. Una mobilitazione allargata in breve tempo su scala nazionale, anche attraverso l'aiuto di giornali, TV, Internet, con raccolte di fondi e catene di solidarietà volte a risolvere l'emergenza sangue e a fornire beni di prima necessità ai rifugiati, con la nascita di punti di raccolta spontanei nelle varie città italiane, a testimonianza della vera identità di un Paese e a dispetto di chi ci dipinge sempre in maniera caricaturale. Ribadiamo il nostro appoggio al Governo per tutte le iniziative che vorrà mettere e che ha già messo in atto per far fronte all'emergenza e apprezziamo gli sforzi che fin qui ha profuso. a proposito di iniziative istituzionali, siamo felici di aderire fin da subito e con entusiasmo, signor Presidente, anche alla sua iniziativa di una sottoscrizione aperta a tutti i soggetti del Senato, parlamentari ma anche dipendenti, a favore delle vittime di questo terremoto. Anche noi ringraziamo i colleghi senatori a vita Ciampi e Colombo per la particolare generosità dimostrata e personalmente dichiaro la mia disponibilità a devolvere l'indennità parlamentare di aprile in favore delle vittime del terremoto. Di particolare rilevanza ci è parsa inoltre la generosità dimostrata da molti Paesi esteri nei confronti dell'Italia i quali hanno messo a disposizione fin da subito aiuti ed esperienza accumulata in tanti interventi di emergenza di questo tipo; ausili di cui il Governo per ora ha deciso, come è nel suo pieno diritto, di non avvalersi, ad eccezione di quelli offerti dagli Stati Uniti. La reazione degli italiani, uniti e solidali di fronte alla sventura di tanti loro connazionali, è stata quindi accompagnata da una politica responsabile e davvero a fianco dei cittadini. Per una volta sono cessate le sterili polemiche e si è riscoperta quella unità di intenti tra maggioranza e opposizione che servirebbe davvero al Paese in questa fase di crisi economica. Si è detto: la tragedia in Abruzzo si poteva evitare. Ma di fronte al susseguirsi degli avvenimenti, alla grave emergenza, si è data giusta precedenza alle soluzioni immediate, convinti che arriverà, e guai se non arrivasse, il tempo di accertare le eventuali responsabilità. Colleghi senatori, quando la natura colpisce con questa forza d'urto sembra che all'uomo non resti che arginare e limitare i danni. Ma tragedie come quelle avvenute in Abruzzo e prima ancora nel Belice, in Umbria, in Molise, in Irpinia, solo per citare le più recenti, ci ricordano che spesso imperizie e negligenze hanno reso ancor più grave il bilancio delle vittime. Innanzitutto, occorre adeguare le abitazioni a standard di sicurezza antisismici, fin dal prossimo piano casa. Sappiamo che su questo tema l'Italia è in netto ritardo, come sappiamo che c'è già la volontà del Governo di intervenire in questo senso. Le nostre regole antisismiche vivono di proroghe dal 2005 e, secondo recenti stime, in Italia ci sono circa 80.000 edifici pubblici da consolidare e 9.000 scuole situate in aree a rischio e realizzate senza criteri antisismici. In totale, poi, il 65 per cento delle abitazioni civili della Penisola risulta poco sicuro. Né abbiamo la certezza che gli edifici costruiti con criteri antisismici siano davvero sicuri in caso di terremoto. All'Aquila ne abbiamo avuto, purtroppo, una triste dimostrazione: abitazioni ed importanti strutture pubbliche sono collassate con sconcertante facilità di fronte al terremoto, segno che le misure finora adottate per la messa in sicurezza degli edifici non sono bastate ad evitare violazioni e truffe nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni comunali di cui solo oggi viene pagato il drammatico prezzo. Bisogna accertare anche penalmente le responsabilità di imprese, progettisti, collaudatori, tecnici ed amministratori che hanno consentito la realizzazione di opere non a norma. All'adeguamento dell'edilizia a reali criteri antisismici deve poi seguire il costante potenziamento e l'aggiornamento delle tecniche di monitoraggio per tentare di prevedere e, quindi, eventualmente limitare i danni in caso di calamità naturali. Bisognerà poi impegnarsi attivamente per ricostruire laddove una catastrofe ha distrutto, per permettere alla popolazione di ripartire e di non vivere perennemente nello *status* di terremotati. Quando si spegneranno le luci delle telecamere, infatti, non siamo certi che tutti continueranno a dimostrare la stessa solidarietà promessa e che molti problemi per gli sfollati non resteranno irrisolti. Non si può pensare che le persone possano essere condannate a vivere tutto il resto della loro vita in *container*, per quanto molto più accoglienti e a norma delle baracche. Bisogna, insomma, evitare che i sopravvissuti ad un terremoto debbano vivere condizionati da questa esperienza per sempre, nella vita di tutti i giorni, oltre che nel ricordo. Nell'Abruzzo il terremoto non solo ha raso al suolo città, ma ha reso irreversibile la già grave crisi economica ed occupazionale. Noi dobbiamo lavorare non solo per la completa ricostruzione: dobbiamo lavorare per ricostruire anche un nuovo e virtuoso sistema economico che rilanci lo sviluppo di quei territori. Signor Presidente, cari colleghi, anche da un evento drammatico come il terremoto in Abruzzo si possono ricavare segnali e spunti di positività. Su tutti, una ritrovata coesione nazionale, a partire dai cittadini, certo, ma anche da una politica che è tornata in qualche modo ad avvicinarsi alla gente. Quando la politica si occupa di cose concrete, non si perde in un bicchier d'acqua e capisce la differenza tra la polemica inutile ed il momento in cui si deve lavorare in concordia, solo allora ritrova un legame con i cittadini. Signor Presidente, colleghi senatori, ora è il momento della responsabilità e della solidarietà nazionale per le popolazioni dell'Abruzzo, così duramente colpite da questo terremoto. Impegniamoci tutti, con serietà e senza troppe parole. Sperando che, una volta passata l'emergenza, non si debba aspettare un altro dramma per ritrovare lo spirito costruttivo di questi giorni.

che l'intero Senato ha inteso assumere nei confronti della mia Regione, l'Abruzzo. Credo che il dovere primario di tutti noi in questo momento sia soprattutto far uscire dall'emergenza le popolazioni dell'Aquila e dei Comuni vicini. Dobbiamo assistere i superstiti, aiutare le famiglie delle vittime,

per un dramma psicologico, all'interno delle auto. Ringrazio il ministro Vito che, a nome del Governo, è venuto a riferire al Senato una nota informativa che è estremamente dettagliata nei numeri e nelle misure assunte. Però, signor Ministro, non c'è nessuna nota informativa che riesca a dare un quadro completo e realistico del dolore e della disperazione che in questo momento stanno vivendo le nostre popolazioni. Bisogna vedere per poter credere: L'Aquila è una città devastata e bombardata dalla violenza della natura. L'Aquila è una città fantasma e di sfollati. I numeri che lei ha dato, signor Ministro, vanno rapportati alla realtà della città.

In quel comprensorio territoriale vi sono 3.000 persone che hanno già perso il lavoro e che ora hanno perso anche la casa.

chiuso i battenti intere grandi industrie. Quando lunedì, alle ore 20, sono andato via dall'Aquila, dopo aver camminato per diverse ore lungo questa città devastata, ho lasciato i soccorritori che ancora stavano scavando con le mani nella speranza di riuscire a tirar fuori dalle macerie gli studenti che erano seppelliti nella Casa dello studente e lungo il viaggio di ritorno ho incrociato code di autoveicoli e mezzi di soccorso. Questi sono per noi abruzzesi due esempi, signor Ministro, di straordinaria solidarietà.

uno straordinario esempio di solidarietà e di coesione sociale, espressione che in passato in questo Paese è rimasta troppo spesso vuota e che ora riusciamo a tradurre in sostanza con atti concreti che vengono assunti nei confronti della nostra Regione.

per quali ragioni quelli che dovevano essere i baluardi della sicurezza per i cittadini più deboli, per i giovani, per le persone che avevano bisogno in un momento drammatico di un punto di riferimento, quei baluardi che dovevano essere l'ospedale, la prefettura,

le morti che forse potevano essere evitate, il nostro Paese ha bisogno di un grande piano di prevenzione, ha bisogno di un imponente progetto di pianificazione per mettere a norma gli edifici pubblici che rappresentano la ricchezza del nostro Paese.

in terremoto. L'impegno futuro del Parlamento sarà quello di vigilare attentamente sulla ricostruzione, perché gli esempi del passato non ci confortano, non ci aiutano. Il Paese ha speso 140 miliardi dal dramma del Belice ai terremoti successivi dell'Irpinia, del Molise, dell'Umbria, delle Marche,

massima trasparenza, rigore amministrativo, tempestività negli interventi. Andando via dall'Aquila siamo stati avvicinati da alcuni cittadini, signor Ministro, ci hanno rivolto un appello che io trasmetto, così come mi è stato lanciato, all'intera Assemblea. Ci hanno detto: non ci lasciate soli dopo. Non in questo momento, in cui la solidarietà è forte: non ci lasciate soli dopo. E noi su questo dopo, signor Ministro, faremo il nostro dovere vigilando e intervenendo affinché le istituzioni possano essere vicine al Paese.

innanzitutto voglio esprimere la vicinanza del Gruppo dei senatori della Lega Nord ai familiari delle vittime del disastro dell'Abruzzo. Di fronte a catastrofi come questa le uniche regole possibili sono silenzio e rispetto. Il silenzio, perché davanti alla morte le polemiche si riducono ad una mera azione di sciacallaggio. Il rispetto, perché è l'unico atteggiamento accettabile di fronte a chi ha perso in modo così traumatico i propri cari e le proprie cose. La Lega Nord è con quei tantissimi cittadini che si stanno adoperando per lenire le sofferenze di queste popolazioni tanto dolorosamente colpite. È un fatto che, non appena apprese le proporzioni del disastro abruzzese, la mobilitazione è stata generale. Moltissime persone, animate solo da grande spirito di solidarietà, insieme ad associazioni, istituzioni, enti locali, tutti si sono messi a disposizione per aiutare le popolazioni colpite dal sisma, chi inviando viveri, chi recandosi sul posto di persona, chi donando sangue o denaro. Davvero un grande slancio di generosità. E per questo voglio ringraziare, insieme alla Protezione civile e ai tanti volontari (non solo del nostro Paese), tutte le forze dell'ordine (Polizia, Carabinieri, Corpo forestale dello Stato, Guardia di finanza, Esercito, i nostri Alpini), chi presta servizio nella sanità a tutti i livelli (amministratori, sindaci, presidenti, assessori e consiglieri di maggioranza e opposizione di tutti i Comuni, Province e Regioni). Tutti in questo momento si stanno muovendo per alleviare le sofferenze delle popolazioni dell'Abruzzo. Intervengo io, a nome del mio Gruppo, in quanto vengo dal Friuli, la Regione padana che, per averlo provato sulla propria pelle, ha un'idea ben chiara della portata del dramma che si sta vivendo in quelle zone. Il 6 maggio del 1976 ero tra coloro che hanno vissuto in prima persona l'incubo di quel tremendo minuto di furia della natura, che sembrava non finire mai. Un rumore crescente fino a diventare assordante, nel buio più totale, con la netta sensazione che l'abitazione stesse crollando, anche se nel mio caso, per fortuna, non è stato così. Memore di quell'esperienza, lunedì, appena dall'Abruzzo sono arrivate le prime notizie, tutto il Nord insieme al resto del Paese si è mosso con volontari, Vigili del fuoco, unità cinofile e tecnici attrezzati di mezzi motorizzati, cucine da campo, ambulanze e fuoristrada, come le popolazioni della nostra penisola sanno fare nei momenti davvero duri. Ed è qui che si misura la forza di un Paese. Se si sanno individuare obiettivi comuni e ci si muove nella stessa direzione, si vince. Come Lega Nord ci stiamo battendo, cercando di coinvolgere anche le altre forze politiche per arrivare a uno Stato federale, dove a tutti i livelli chi amministra è responsabile delle proprie azioni e quindi ne risponde. In passato, forse, non c'è stata particolare attenzione alla prevenzione. Ecco, per il futuro sarà un nostro preciso impegno vigilare sul rispetto delle regole. Ogni opera, pubblica o privata che sia, deve avere ben chiaro il nome di chi ne è responsabile. Per intanto siamo soddisfatti di come in questa emergenza si sta muovendo il Governo e, in particolare, il nostro Roberto Maroni, Ministro dell'interno, che ha fornito i primi numeri dell'emergenza. Già il primo giorno, nel giro di poche ore, erano confluiti per prestare soccorso all'Aquila, da varie parti del Paese, 1.500 vigili del fuoco, centinaia di poliziotti e carabinieri. Gli sfollati vengono sistemati in alberghi e in strutture già costruite o in corso di costruzione. La situazione, insomma, è sotto controllo. Fanno la loro parte - lasciatecelo ricordare - anche le associazioni vicine al nostro movimento, non solo provenienti dal Nord, ma anche dai territori prossimi alle zone colpite. Ne andiamo fieri. Verrà poi il momento di quantificare i danni. Sono già stati stanziati per i provvedimenti più urgenti 30 milioni di euro. Domani, in Consiglio dei ministri, con un quadro più chiaro sia per quanto riguarda la portata del disastro sia sulla disponibilità di risorse strutturali, si parlerà concretamente delle cifre da mettere a disposizione. Per la ricostruzione degli edifici il modello ideale cui ispirarsi è forse proprio quello del Friuli, dopo il terremoto del 1976, caratterizzato da una particolare unitarietà di obiettivi fra le diverse parti in causa. Unità d'intenti culminata con l'emanazione - avvenuta solo 7 giorni dopo il sisma - del decreto-legge che ha permesso ai Comuni di scegliere autonomamente quali operazioni attuare per la ricostruzione territoriale, sapendo di avere alle spalle istituzioni come Regione e Governo pronte a condividere le scelte. Grazie a un'attenta e oculata gestione delle risorse, dopo soli dieci anni i Comuni più colpiti erano già ricostruiti. Come già annunciato dal Presidente del nostro Gruppo, Federico Bricolo, i senatori della Lega Nord aderiscono all'iniziativa del presidente Schifani per una raccolta di fondi a sostegno delle famiglie colpite dal sisma. Riteniamo infatti che mai come in questo momento sia giusto dare un segnale concreto di solidarietà a chi sta soffrendo. *(Applausi

anche rispetto alla storia recente del rapporto tra le istituzioni e le situazioni di difficoltà che si sono verificate nel nostro Paese.

dopo le giornate passate, la vicenda vissuta, c'è nervosismo anche in una popolazione come questa, che è particolarmente sobria e forte.

sia per l'estensione del patrimonio verde e montano, sia per la storia che ha conosciuto, per i reperti architettonici, culturali, religiosi, insomma per la civiltà.

La grande speranza di questo polo industriale che si è insediato nel Fucino, ad Avezzano, la Micron, ha conosciuto la cassa integrazione, che è stato un duro colpo per le popolazioni

quattro anni) come a una ricchezza, a un patrimonio dell'Europa, e più vengono più si confermano in questa posizione.

La prospettiva è quella di non abbandonare il recupero del valore del territorio. Caro senatore Piccone, in quella zona c'è una prospettiva anche agricola, ma il suo centro è inserito in un percorso storico, artistico e culturale straordinario. la capitale della Lega italica, dell'ultima resistenza ai romani, era nel cuore di questo territorio. Oggi è un piccolissimo paese vicino a Sulmona: si chiama Corfinio.

Signor Presidente, colleghi senatori, signori rappresentanti del Governo, permettetemi in primo luogo di ringraziare lei, Presidente, per le belle parole e la sensibilità dimostrata nei confronti del nostro dramma; i colleghi che mi hanno preceduto e, soprattutto, il presidente Marini che ha avuto parole di grande affetto e che, dall'alto della sua onestà intellettuale e politica, ha saputo riconoscere, in un momento come questo, anche dai banchi dell'opposizione, ciò che il Governo sta mettendo in campo. È con grande tristezza che mi accingo a svolgere il mio intervento, sentendo la responsabilità di parlare a nome del Gruppo del PdL, io, abruzzese e cittadino aquilano. La gravità dell'evento che ha drammaticamente colpito l'Abruzzo, la mia Regione, m'induce a parlare in quest'Aula, nonostante il profondo dolore che provo per le vittime, i loro familiari e per l'intera comunità abruzzese. L'intervento del rappresentante del Governo è stato chiaro e analitico e, pur nella doverosa laconicità dei dati, ha lasciato trasparire, da un lato, la percezione del dramma, dall'altro, il senso di uno Stato pronto ad intervenire con tempi rapidi e progetti chiari. Voglio esprimere la mia e la nostra vicinanza alle popolazioni colpite, il nostro affetto umano, il nostro più forte senso di solidarietà. Desidero, inoltre, subito tributare la nostra profonda gratitudine a tutti coloro che da giorni si stanno prodigando per soccorrere le popolazioni terremotate. Mi riferisco agli straordinari volontari abruzzesi e di ogni parte d'Italia, alla Protezione civile, ai Vigili del fuoco, alla Croce rossa, al sistema sanitario, alle forze dell'ordine e alle In uno scenario apocalittico, la macchina dello Stato ha operato con prontezza ed efficienza, garantendo soccorsi immediati attraverso i suoi bracci operativi, soccorsi che ogni ora si dimostrano, oltre che vitali, basati su altissima professionalità e, al tempo stesso, permeati di straordinaria umanità: tutto ciò, quasi a lenire - come fosse possibile - il senso del dolore o dello smarrimento che si sta vivendo. Una grande solidarietà alle vittime del terremoto ha animato le istituzioni, i volontari e le singole persone. A fronte della più grande tragedia del nuovo secolo per il nostro Paese, è tornato ancora una volta a pulsare il grande cuore degli italiani, unitamente alla loro grande operosità. Su questo, per inciso, vorrei esprimere un attestato di gratitudine particolare a voi, colleghi senatori, e agli onorevoli deputati, per le sottoscrizioni avviate dai presidenti Schifani e Fini, che hanno subito raccolto il consenso unanime e *bipartisan* dei parlamentari di tutti gli schieramenti politici. La tragedia che ha colpito la mia Regione ha posto l'intera classe politica di fronte alle proprie responsabilità. Posso affermare che il confronto politico in questa occasione ha riacquistato dignità grazie al buonsenso e alla disponibilità manifestati da tutti gli schieramenti, restituendo alla politica quel senso di nobiltà che spesso perde e dimostrando che il nostro compito primario resta quello di affrontare i problemi. La drammaticità dell'evento ha generato un nuovo senso di coesione nazionale, che da giorni permea il dibattito politico: una linea responsabile, basata sul rispetto reciproco, ha caratterizzato il confronto tra Governo e opposizione. E infatti, anche la discussione odierna sta delineando un nuovo scenario, nel quale le posizioni propositive e collaborative hanno dato forma ad un dibattito politico responsabile, dignitoso ed efficace. In questo contesto, assume un significato importante ed alto la presenza del Presidente del Consiglio Il suo impegno diretto rappresenta per tutti noi una testimonianza molto forte, che da subito ha segnato la presenza dello Stato, del Governo e di tutta la classe dirigente del Paese. Il Governo - posso dirlo con cognizione di causa - ha dato e sta dando in queste ore agli abruzzesi parole di speranza e certezza nel futuro. Gli impegni assunti in termini di assistenza immediata, ma soprattutto la progettualità tecnica ed economica che il Governo ed il presidente Berlusconi hanno già messo in campo, può farci dire che ci attende una grande sfida che siamo pronti a vincere tutti assieme, con assoluta rapidità. Questa è la promessa Questa è la promessa solenne che oggi dal Senato della Repubblica rivolgiamo alle donne e agli uomini d'Abruzzo, così ingiustamente e ferocemente colpiti. Il mondo intero osserva commosso il composto dolore del popolo abruzzese, che nell'affrontare una tragedia di tale portata sta dimostrando lucidità, sobrietà, pudore e determinazione. L'immagine di una Regione che negli ultimi mesi era risultata appannata sta invece dimostrando il suo volto migliore, quello di chi a volte cade, ma poi sempre si rialza e riprende il cammino. L'Abruzzo si sta proponendo come una Regione laboriosa anche in quest'occasione: riuscirà, avendone i mezzi, le risorse e la volontà, a superare la crisi. Sappiamo che ciascuno di tali elementi è già messo a disposizione: la nostra grande responsabilità sarà quella di saperli fondere per utilizzarli subito e bene. Il nostro cuore in ogni momento è in Abruzzo. Le nostre capacità, in quest'Aula, secondo le competenze di ciascuno, sono e saranno, da oggi ancora di più, al servizio vero dei cittadini: possiamo e vogliamo farlo. Ricostruire L'Aquila, le sue mura, i suoi monumenti, le sue scuole e il suo intero tessuto sociale ed economico sarà una missione prioritaria: con determinazione e senso civico lo faremo, presto e bene. Questo è il compito delle istituzioni, questo è l'obiettivo di noi tutti: sarà il modo migliore e più utile di stringere gli abruzzesi e tutti gli italiani in un unico, intenso abbraccio, per guidarli verso una rinascita per l'oggi e per il futuro*.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1503 prevede la conversione in legge del decreto-legge n. 5 del 2009, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. Il provvedimento, approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, è stato esaminato delle Commissioni riunite 6a e 10a. Tra le misure di maggiore interesse per l'industria italiana si segnalano le previsioni contenute nell'articolo 1, con il quale sono stati introdotti dei significativi incentivi per il rinnovo del parco auto, nonché per l'acquisto di veicoli ecologici. In particolare, nei commi da 1 a 10 dell'articolo 1 è prevista la concessione di incentivi per la rottamazione di veicoli inquinanti, per l'acquisto di veicoli ecologici e per l'installazione di impianti a metano o a GPL. Un contributo di 1.500 euro è previsto per l'acquisto di autovetture Euro 4 o Euro 5, in sostituzione di auto immatricolate entro il 31 dicembre 1999, di categoria Euro 0, Euro 1 o Euro 2. Un ulteriore contributo pari a 1.500 euro è previsto per l'acquisto di auto a GPL; il contributo è invece di 3.500 euro per le autovetture alimentate a metano. Gli incentivi per le rottamazioni sono altresì previsti per i veicoli commerciali e per l'acquisto di nuovi motocicli Euro 3 a fronte della rottamazione di un ciclomotore Euro 0 o Euro 1. L'articolo 3 reca una serie di misure a favore dei distretti produttivi e delle reti di impresa, attraverso uno specifico intervento sulla disciplina fiscale dei distretti produttivi. A tale proposito ricordo che delle disposizioni di analogo contenuto sono presenti anche nel disegno di legge n. 1195 all'esame della Commissione industria del Senato. Si segnala inoltre che l'articolo 3, ai commi 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies*, prevede la disciplina del contratto di rete, che può essere stipulato da due o più imprese che si obbligano ad esercitare in comune L'articolo 4, nei commi da 1 a 7, introduce una serie di disposizioni volte a favorire le aggregazioni di imprese effettuate nell'anno in corso attraverso operazioni di di fusione e scissione. Per raggiungere questo obiettivo si permette il riconoscimento fiscale gratuito del valore maggiore attribuito ai beni materiali e immateriali. Tali misure, pertanto, si collocano nella scia già delineata dalla Commissione industria del Senato con l'approvazione della risoluzione nell'ambito dell'esame dell'Atto comunitario n. 8, meglio noto come *Small business act*. L'articolo 4, al comma 7-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede inoltre una dotazione di 300 milioni di euro a sostegno del credito per favorire le esportazioni di prodotti *made in Italy*. L'articolo 5-*bis*, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati, introduce delle norme finalizzate a favorire la riconversione degli impianti industriali di energia elettrica ad olio combustibile, al fine di permettere l'alimentazione a carbone o ad altro combustibile solido. L'articolo in esame prevede sostanzialmente una deroga ai limiti di localizzazione degli impianti previsti dalla normativa nazionale e da quella regionale. L'articolo 6, al comma 1, introduce l'intervento della SACE S.p.A. per la prestazione di idonee garanzie al fine di agevolare l'erogazione dei finanziamenti volti all'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli commerciali destinatari degli incentivi previsti dall'articolo 1 del provvedimento d'urgenza. 7, al comma 1-*quinquies* e 1-*sexies*, al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, anche in considerazione dell'attuale crisi economica internazionale, prevede degli interventi a sostegno di imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature. In particolare nel comma 1-*quinquies* è previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro al fine di fornire delle garanzie, anche mediante ricorso ai consorzi di garanzia fidi, alle imprese operanti nei distretti produttivi nel settore della concia, del tessile e delle calzature. Nell'ambito dell'articolo 7, invece, è prevista una serie di misure di semplificazione e realizzazione delle procedure inerenti gli ammortizzatori sociali. In particolare, tra gli interventi previsti, si segnala l'autorizzazione del pagamento diretto da parte dell'INPS dell'indennità contestualmente all'autorizzazione del trattamento di cassa integrazione. Gli articoli 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, infine, prevedono una serie di disposizioni in materia di quote latte. Da ultimo vorrei segnalare che, nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite, è stato approvato un apposito ordine del giorno che impegna il Governo ad inserire in un prossimo provvedimento legislativo una moratoria per la riscossione dei canoni demaniali per le concessioni relative agli stabilimenti balneari. Si tratta di un atto importante e significativo di supporto non solo al settore commerciale e industriale ma anche a quello rilevante del turismo, anch'esso in crisi per le note vicende. Tale problematica, affrontata nel corso dell'esame del provvedimento d'urgenza da parte della Camera dei deputati, non ha poi trovato una compiuta soluzione. Risulta pertanto auspicabile che il Governo, anche alla luce dell'ordine del giorno approvato dalle Commissioni riunite all'unanimità, fornisca in tempi rapidi una soluzione a questo problema che coinvolge numerosi operatori di un settore strategico per l'economia nazionale come quello del comparto turistico-balneare.

Signor Presidente, il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. al cui interno è stato anche inglobato il testo del decreto-legge n. 4 del 2009 m materia di quote latte, reca un contenuto che incide su ambiti normativi differenziati, con misure tuttavia accomunate, nelle intenzioni del Governo, dall'esigenza di fronteggiare le ripercussioni dell'attuale crisi economico-finanziaria su più fronti. Relativamente alle parti di competenza della 6a Commissione, intendo segnalare sinteticamente le seguenti disposizioni. L'articolo 2 prevede una detrazione del 20 per cento delle spese documentate, nella misura massima di 10.000 euro ripartita in cinque annualità, sostenute per l'acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo di un immobile per il quale siano effettuati interventi di ristrutturazione edilizia. L'articolo 3, commi da 1 a 3 e comma 4, modifica la disciplina fiscale dei distretti produttivi, estesa anche alle reti di imprese e alle catene dì fornitura, reintroducendo il regime fiscale previsto dalla legge finanziaria 2006 (disciplina che non aveva trovato applicazione in mancanza dei relativi decreti attuativi), prevedendo la facoltà di optare per il regime della tassazione consolidata di distretto o per la tassazione preventiva concordata triennale. I commi 3*-bis* e 3*-ter* prevedono poi che le agevolazioni previste per la sostituzione di veicoli, di mobili ed elettrodomestici si applicano solo nei confronti delle aziende che si impegnano a non delocalizzare la produzione al di fuori dello Spazio economico europeo. Il comma 4*-bis* amplia la tipologia delle diverse forme di finanziamento che possono essere effettuate nell'ambito della gestione separata della cassa depositi e prestiti. L'articolo 3*-bis* prevede la possibilità di estendere il regime IVA ad esigibilità differita, di cui all'articolo 7 del decreto-legge

L'articolo 4, commi da 1 a 7, introduce un beneficio fiscale diretto a favorire le aggregazioni aziendali (fusione, scissione e conferimenti) effettuate nel 2009 attraverso il riconoscimento gratuito del maggior valore attribuito ai beni materiali e immateriali cui corrisponde, per le fusioni e le scissioni, una differenza da concambio. L'agevolazione spetta entro il limite massimo di maggior valore pari a 5 milioni di euro. L'articolo 5, al comma 1, provvede a ridurre le aliquote dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione ed il riallineamento volontario dei valori contabili degli immobili non merce dal 7 al 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dal 4 all'1,5 per cento per quelli non ammortizzabili. L'articolo 7 reca norme in materia di potenziamento dei controlli fiscali e di inasprimento delle sanzioni per l'indebito utilizzo di crediti in compensazione. Viene prevista una forma di controllo mirato sulle agevolazioni previste per alcune imposte indirette (registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni); si incrementano di 4 milioni di euro gli stanziamenti per gli anni 2009 e 2010 per l'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale; si prevede una sanzione del 200 per cento dell'importo corrispondente al credito indebitamente compensato per tutte le ipotesi in cui siano state effettuate compensazioni con crediti inesistenti per importi superiori a 50.000 euro; si prorogano i termini per l'esecuzione delle procedure di recupero degli aiuti di stato indebitamente percepiti dalle società cosiddette ex-municipalizzate. Significative le modifiche apportate con i commi 3-*quater*, 3-*quinquies* e 3-*sexies* in materia di mercati finanziari, in virtù delle quali viene aumentata la misura della quota di partecipazione che l'azionista di controllo può incrementare senza che sia soggetto all'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria, viene affidata alla CONSOB la facoltà di ridurre al di sotto del 2 la soglia per le comunicazioni delle partecipazioni rilevanti, e viene aumentata la misura (dal 10 al 20 per cento) delle azioni proprie che possono essere acquistate. L'articolo 7-*quater* reca disposizioni in materia di Patto di stabilità interno dirette sostanzialmente a ridurne i vincoli relativamente alle spese di investimento. Si escludono dal computo del saldo utile ai fini del Patto per l'anno 2009 determinate tipologie di spese in conto capitale, nonché le spese per interventi temporanei e straordinari di carattere sociale a favore di lavoratori e imprese (limitatamente ai soli enti locali virtuosi); per le Regioni che rendono disponibili gli importi necessari a garantire la spesa degli enti locali nel 2009, è autorizzato lo svincolo di destinazione di somme ad esse spettanti, provenienti da trasferimenti statali per un importo pari al doppio degli importi resi disponibili; vengono stanziate ulteriori risorse per l'avvio di interventi di edilizia residenziale pubblica; per le Regioni, a decorrere dal 2009 vengono escluse le spese correnti per interventi realizzati con cofinanziamenti dell'Unione Europea, per la sola parte di finanziamento europeo, dal computo delle spese considerate ai fini del rispetto del Patto di stabilità. L'articolo 7-*octies* è infine finalizzato al rimborso dei titolari di obbligazioni emesse dalla società Alitalia, attualmente in amministrazione straordinaria. In particolare, la disposizione si applica ai titolari delle obbligazioni "Alitalia

apre una nuova finestra"), *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni: in relazione all'articolo 7, con particolare riferimento al comma 1-*bis*, il meccanismo contabile delineato tiene conto delle specifiche procedure di ripartizione delle risorse e risulta scontato nei tendenziali di spesa a legislazione vigente; in relazione all'articolo 7-*quater*, pur non risultando specificati i meccanismi di salvaguardia, restano comunque fermi gli obiettivi programmati in materia di Patto di stabilità interno; in relazione all'articolo 7-*quinquies* la destinazione delle risorse tiene conto della diversità degli interventi da finanziare, sia di natura corrente sia di parte capitale, la cui natura potrà essere specificata solo al momento della ripartizione del fondo stesso. Il parere è altresì reso nel presupposto che: con riferimento all'articolo 3, l'amministrazione operi secondo le modalità successivamente definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel rispetto del vincolo finanziario di cui al comma 4; con riferimento all'articolo 4, il valore relativo ai beni strumentali e immateriali non ricomprenda quello relativo all'avviamento; con riferimento all'articolo 6, nei confronti delle operazioni poste in essere dalla SACE S.p.A., non operi la garanzia dello Stato di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 269 del 2003; con riferimento all'articolo 7-*octies* risultino disponibili le risorse di cui all'articolo 1, commi 343 e 345, legge n. 266 del 2005, relativo ai cosiddetti conti dormienti». Presidente, in considerazione della ravvicinata data di scadenza del decreto-legge e della particolare importanza che il Governo attribuisce alla tempestiva approvazione delle norme ivi contenute, così come testé illustrate dai relatori, che ringrazio, a nome

Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi senatori, la notizia che adesso il Governo ha ufficializzato, circa la volontà di porre la questione di fiducia a questo disegno di legge, riduce chiaramente lo spazio e la virtuosità del nostro dibattito. Ciascuno di noi è chiamato a questo punto a fissare alcune posizioni che servano a rendere chiaro il quadro delle responsabilità e il senso degli indirizzi generali. Questo provvedimento, che nasce per

è diventato, come spesso avviene nell'*iter* parlamentare, qualcosa di molto diverso: è ormai un assemblaggio di diverse proposte, indicazioni, suggestioni, incentivi ed altro. Ci dobbiamo porre il problema se deve essere questo il modo in cui il sistema Paese guarda alle istituzioni con fiducia e serenità e se è questo il modo per uscire dalla crisi

la fiducia di cui l'economia ha bisogno. Signori del Governo, colleghi senatori, quando la crisi diventa acuta e quando il sistema si "imballa", in genere si pensa di riattivarlo attraverso un'incentivazione del ruolo, della funzione e della responsabilità degli enti locali. Recentemente, un grande commentatore, lucido come sempre, Eugenio Scalfari, l'ha ricordato a noi tutti e credo che sia giusto rammentarlo perché non è una questione che possa dividere il Parlamento tra chi è favorevole e chi è contrario, ma è una scelta che in genere corrisponde all'interesse generale del Paese. Cosa c'è per riattivare il volano dell'economia locale secondo una funzione attiva degli enti locali? Pochissimo, veramente poco. Recentemente l'Associazione nazionale dei Comuni italiani ha ricordato che sono impigliati nei bilanci comunali circa tre miliardi di avanzi di amministrazione e circa 15 miliardi di residui passivi. Sono risorse che potrebbero essere destinate ad un processo necessario, quello della riattivazione della nostra economia, operando più investimenti, realizzando più opere pubbliche, riattivando e rilanciando la macchina della nostra attività produttiva locale. Eppure, nel provvedimento in questione - il relatore ne ha accennato fugacemente ed in maniera poco chiara - c'è davvero una misura che contraddice questo spirito e questa volontà. È vero, si stabilisce che i Comuni virtuosi possono riaprire parzialmente i cordoni della spesa, e derogare parzialmente al Patto di stabilità. Questa opportunità, però, è circondata da un eccesso di cautele e, soprattutto, cari colleghi, si accompagna ad una misura che suona come una beffa. Infatti, nel giro di pochi giorni, entro il mese di maggio, quando le Regioni già avranno chiuso i loro bilanci, si dovrebbe procedere ad un'operazione rocambolesca:

i frutti e gli esiti della finanza creativa. Il ministro Tremonti sostiene di avere sempre previsto tutto. Quando era Ministro del tesoro nel 2001 ha lasciato che si aprisse questo nuovo corso della finanza creativa; i Comuni hanno dilatato i loro investimenti, hanno prolungato ed allungato il proprio debito, hanno fatto ricorso a tutti i nuovi sistemi di finanziamento. Oggi ci accorgiamo che il debito poca cosa rispetto a quello del sistema Paese - è cresciuto troppo ed allora dobbiamo intervenire. Se fossimo intervenuti prima, mantenendo una posizione di razionalità e di coerenza, oggi non

la discussione che stiamo svolgendo rischia di apparire, per varie ragioni, del tutto surreale. surreale. Infatti, abbiamo perso il conto dei provvedimenti adottati dal Governo per contrastare la crisi, provvedimenti parziali e sempre più inadeguati e drammaticamente in ritardo.

I dati a nostra disposizione mostrano una realtà ogni giorno più drammatica. Alcuni istituti di ricerca hanno elaborato delle analisi che prevedono entro il 2010 oltre un milione di posti di lavoro persi nel triennio, mentre alla fine di questo anno i disoccupati in più sarebbero circa 500.000, con un tasso di disoccupazione che dovrebbe salire a oltre il 9 per cento, e al 10 per cento nel 2010, a fronte del 7,4 per cento Più di questi numeri parlano le file dei cittadini comuni, per lo più anziani, davanti alle mense della Caritas e addirittura gli aumenti dei furti di alimenti nei supermercati. È bene ricordare che, anche per quei lavoratori che sono in cassa integrazione, il rischio di trovarsi nella fascia della povertà è sempre più reale. Gli ultimi dati della cassa integrazione mostrano un aumento superiore al 200 per cento, con picchi del 300 per cento per alcuni comparti produttivi. Le peggiori situazioni investono

Sono sostanzialmente colpite tutte le Regioni italiane. Le 52 settimane di cassa integrazione stanno per esaurirsi; da più parti viene richiesto al Governo di raddoppiarle: sarebbe una cosa giusta e necessaria. Se alcune misure presenti nel decreto sono condivisibili - penso al settore dell'auto - ci domandiamo perché non siano state introdotte prima, in tempo per provare ad interrompere questo disastro.

Sabato scorso si è svolta a Roma una grande manifestazione di lavoratori, di un pezzo del nostro Paese che soffre quotidianamente in prima persona questa crisi. Da quella manifestazione è arrivato un invito al Governo: apriamo un tavolo di confronto, uniamo le forze. A questa richiesta, tutt'altro che evasiva, si è risposto parlando di scampagnate e di tavolini rivoltati. Siamo - lasciatemelo dire - all'irresponsabilità, siamo al contrario di ciò che un Governo dovrebbe fare in questa situazione. Noi, come PD, abbiamo avanzato delle proposte concrete e sostenibili finanziariamente. Penso all'estensione della cassa integrazione, all'assegno di disoccupazione e ancora alla proposta di una moratoria contro il licenziamento per tutto il 2009 dei precari della pubblica amministrazione. proposta che coglie un dramma reale che rischia di investire circa 400.000 lavoratori. Inoltre, abbiamo proposto una tassazione straordinaria per i redditi più alti, a cominciare da quelli dei parlamentari. Abbiamo promosso una battaglia parlamentare che alla Camera ha dato luogo all'approvazione, con il consenso della maggioranza, di una mozione per rendere meno stringente il Patto di stabilità degli enti locali, anche se il giorno dopo tale proposta è stata messa in discussione. Ora ci aspettiamo i fatti. Centinaia di imprese rischiano di chiudere a causa dei mancati pagamenti degli enti locali e dell'inasprimento delle linee di credito degli istituti bancari. Facciamo in modo di evitare di spendere soldi pubblici in ammortizzatori sociali nei casi in cui è lo Stato a chiudere le aziende; e comunque evitiamo che queste aziende chiudano. Il nostro è un pacchetto di proposte concrete, semplici e sostenibili finanziariamente. Il ministro Sacconi ha più volte detto che esistono 32 miliardi per gli ammortizzatori sociali, tra fondi ordinari e straordinari. Non si comprende allora la reticenza del Governo ad assumere le nostre proposte che, tra l'altro, non arriverebbero a costare queste cifre. Se il problema è la copertura, anche a rischio di essere tacciato di demagogia, non posso non ricordarvi che in questo Paese esiste una sacca enorme di evasione fiscale. Sarà il caso di far pagare in Italia solamente i 200.000 contribuenti che dichiarano più di 120.000 euro lordi annui; sarà il caso di far pagare quei signori prima o poi. Lo so, è facile demagogia, ma certo la battaglia all'evasione senza più controllo sugli assegni e la cancellazione dall'elenco dei fornitori oggi sarà più difficile di ieri. Certamente l'aver voluto premiare i produttori di latte che non hanno rispettato le regole, a scapito dei tanti che le hanno rispettate pagando in proprio, non è il modo migliore per inviare un messaggio di serietà al Paese. Alle nostre proposte avete risposto con misure parziali, inadeguate, tardive. Credo che avesse ragione il ministro Tremonti quando pochi giorni fa ha sostenuto che chi non ha saputo prevedere il disastro non può essere in grado di prevedere il futuro. Voi non siete stati in grado di prevedere il disastro, visto che tra le prime azioni assunte dal Governo avete pensato bene di detassare gli straordinari e cancellare l'ICI per le case di lusso, e non potete quindi prevedere il futuro,

*(PD)*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, reca misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. Un provvedimento che, per volontà del Governo, nasce per sostenere i settori industriali che producono auto, mobili, elettrodomestici e per rivedere la disciplina tributaria per i distretti produttivi e l'aggregazione tra imprese, ma che non ha previsto nessuna misura per la crisi del settore agro-alimentare.

Presidente, è che di fronte alla crisi economica internazionale le recenti manovre approvate dal Governo non hanno in nessun caso contemplato le parole «agricoltura» e «pesca». Una spiacevole novità tutta italiana, come dimostra il fatto che i principali Paesi europei hanno adottato manovre anticrisi includendo al loro interno misure specifiche per il rilancio competitivo del comparto. cito soltanto il caso della Francia che ha visto il ministro dell'agricoltura Barnier varare un piano di circa 300 milioni di euro per sostenere i redditi degli agricoltori. Al di là dei paragoni è importante evidenziare che l'agricoltura italiana e il settore lattiero-caseario, nello specifico, affrontano oggi uno scenario fatto di mille difficoltà amplificate dalle deficienze strutturali e organizzative e dalla crisi internazionale. I costi produttivi e gli oneri sociali sono raddoppiati; nell'ultimo anno per l'acquisto dei fattori produttivi sono stati registrati aumenti medi del 7 i prezzi all'origine, dopo una fase di rialzo della prima metà dello scorso anno, sono scesi in media del 7 per cento con punte del 35-50 per cento nel mercato dei cereali; i redditi degli agricoltori, dopo l'aumento registrato nel 2008, sono ovunque in calo; migliaia di posti di lavoro sono a rischio (penso al tabacco, ad esempio) e tantissime imprese agricole, costrette sempre più spesso all'indebitamento, stanno uscendo dal mercato.

Oggi per il rilancio competitivo del comparto agro-alimentare il mantenimento dello *status* *quo* non può più bastare. È necessaria una strategia, che abbia una prospettiva di medio-lungo termine, che sappia attivare interventi strutturali profondi. È su questo che bisogna riflettere. Venendo alle disposizioni contenute nell'articolo 8-*bis* del provvedimento, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, noi del Partito Democratico, come abbiamo ricordato anche ieri in Commissione, non avremmo mai modificato la legge n. del 2003, che all'epoca è stata votata dalle attuali maggioranza ed opposizione e che ha prodotto buoni risultati. Voglio ricordare, signor Presidente, che il Partito Democratico durante l'intero *iter* parlamentare ha voluto seguire un atteggiamento costruttivo dato che responsabilmente siamo tutti interessati a chiudere definitivamente l'annosa vicenda delle quote latte - e condiviso anche da tutte le altre forze di opposizione presenti in Parlamento, a cui si è unito lo sforzo profuso dalla maggior parte delle organizzazioni agricole professionali scese in piazza nel corso delle precedenti settimane, per esprimere, a nome degli allevatori italiani onesti, la totale contrarietà al provvedimento del Governo. Tutto ciò, comunque, ha prodotto dei risultati che ci sentiamo in dovere di rivendicare. Mi riferisco al fatto che oggi siamo tornati a discutere del provvedimento approvato in prima lettura dal Senato, da questa Assemblea, ed al cui interno è inserita, non per volontà del Governo ma solo in seguito ad un parere condizionante della Commissione bilancio, su invito dei senatori del PD, la rinuncia espressa ai contenziosi per i produttori che aderiscono alla rateizzazione del proprio debito. Il ritorno al testo approvato dal Senato ha reso possibile anche la proroga al 31 dicembre 2009 delle agevolazioni contributive agricole nelle zone svantaggiate (Mezzogiorno ed aree svantaggiate del Centro-Nord). È stato infatti sventato il tentativo della Commissione agricoltura della Camera che, attraverso un emendamento, aveva ridotto i tempi di tale importantissima proroga al 30 settembre, portando allo sconcerto molte aziende agricole meridionali. Sempre alla Camera, in seguito ad alcuni emendamenti presentati dai deputati della Lega e successivamente approvati in Commissione agricoltura, si era corso concretamente il rischio di un indebolimento della rinuncia ai contenziosi. Mi riferisco alla disciplina della revoca delle quote e, in particolare, al tentativo strumentale di introdurre il termine "reiterato" nei casi di mancato pagamento delle rate. Anche in questo caso, fortunatamente, la ferma contrarietà di tutti i partiti dell'opposizione, e anche di una parte della maggioranza, e le numerose proteste delle organizzazioni agricole sono riuscite a bloccare l'approvazione del provvedimento. Apprezziamo, infine, l'accoglimento dell'ordine del giorno presentato dai colleghi del Partito Democratico alla Camera sul rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, anche se siamo convinti che i 110 milioni di euro siano insufficienti e che, quantomeno, deve essere garantito da questo Governo quanto è stato fatto in precedenza. E ricordo che le precedenti due finanziarie hanno stanziato

La maggior parte delle proposte di modifica presentate al Senato e alla Camera, sia in Commissione agricoltura sia in Aula, puntualmente non sono state approvate dal Governo. Eppure, si è sempre trattato di emendamenti condivisi dal mondo produttivo e dalla maggioranza ed a volte all'unanimità dalle Regioni italiane. Le nostre - onorevoli colleghi - sono state proposte orientate al miglioramento del testo originario e concepite esclusivamente per tutelare i tantissimi allevatori onesti che nel corso degli anni hanno rispettato le regole ed agito nella legalità. In definitiva, signor Presidente, a coloro i quali hanno continuato a produrre latte ignorando la legge avevamo chiesto semplicemente di pagare gli arretrati delle multe e di rinunciare ai contenziosi intrapresi per l'ottenimento delle nuove quote. Proposte chiare, semplici e all'insegna dell'onestà che, tuttavia, sono state respinte dal Governo che, pur di tutelare gli interessi di pochi allevatori disonesti, ha dovuto proseguire per la sua strada ignorando le proposte dell'opposizione condivise dalle Regioni e dalle organizzazioni professionali che - come ricordavo - sono ritornate in piazza. Sono queste le ragioni per cui oggi, grazie peraltro ad una forzatura regolamentare che rischia di creare un precedente preoccupante per la democrazia del Paese, ci troviamo a discutere di quote-latte all'interno di un provvedimento sulla crisi dei settori industriali

Signor Presidente, mi sarebbe piaciuto se in questo provvedimento avessimo potuto affrontare anche la fase della discussione degli emendamenti

che, come qualche altro collega ha già detto prima di me, non appartengono alla maggioranza o all'opposizione, ma appartengono al Paese e che quindi meriterebbero una discussione approfondita, non solo sulle proposte che vengono dal Governo, ma anche sulle proposte che, attraverso gli emendamenti, vengono fatte dall'opposizione.

quello delle piccole e medie imprese. Dico questo perché è indubbio che il nostro sistema imprenditoriale si è storicamente sviluppato intorno ad un gruppo nutrito di grandi imprese operanti in settori strategici e ad alta intensità di capitale, ma anche intorno ad un mondo, ad un'ampia platea di piccole e piccolissime imprese a loro volta attive soprattutto nei cosiddetti settori tradizionali del*made in Italy*. L'equilibrio tra le due dimensioni aveva in passato assicurato la possibilità di mantenere ed accrescere la nostra competitività; alla progressiva fuoriuscita delle grandi imprese nel corso dei passati decenni ha invece corrisposto la tenuta ed il consolidamento del sistema di piccole e medie imprese. In tale scenario non è risultato marginale il ruolo dei distretti industriali. Il nostro tessuto produttivo è così riuscito anche in anni recenti a superare, senza subire impatti particolarmente devastanti, le fasi cicliche avverse. Ricordo che in un sistema imprenditoriale europeo caratterizzato da una larga prevalenza di piccole e medie imprese, l'Italia si distingue per una particolare diffusione della dimensione micro delle imprese.

a poco più della metà degli addetti complessivi, a fronte di quote molto più contenute per tutti gli altri principali Paesi europei. Inoltre, a differenza di quanto avvenuto negli altri Paesi europei, l'Italia ha accentuato il proprio modello di specializzazione, sbilanciato versi i settori tradizionali, in cui è relativamente minore l'importanza dell'economia di scala. Quindi, lo ripeto, la prevalenza di piccole e piccolissime imprese si è consolidata a fronte di una crescita contenuta, per esempio, dei Ecco perché mi sarebbe piaciuto che su questo mondo, che rappresenta la maggior parte del nostro tessuto produttivo, si fosse intervenuti in maniera più incisiva. anche perché, lo ricordava il relatore Cursi, presidente della 10a Commissione, è ormai da un anno che in Commissione attività produttive discutiamo e ci interroghiamo, approvando anche documenti in modo unitario, in ordine alle piccole e medie imprese e poi ci ritroviamo ad approvare provvedimenti legislativi che in realtà incidono in misura assolutamente insufficiente su tale settore. La globalizzazione dell'economia ha contribuito ad un rapido diffondersi della crisi congiunturale. In questa fase recessiva,

Tale debolezza emerge anche in relazione alla dinamica degli incagli rispetto ai prestiti: anche in questo caso il disagio nel rimborso dei prestiti appare più gravoso proprio per le piccole e medie imprese. aumenta il numero delle imprese che si sono viste rifiutare la richiesta di affidamento con una restrizione che, anche in questo caso, sembra colpire soprattutto le piccole e medie imprese. Non parlo poi dell'inasprimento dei criteri applicati per l'approvazione di prestiti e l'apertura di linee di credito a favore, per l'87,5 per cento dei casi, delle piccole imprese. L'irrigidimento riguarda soprattutto l'ammontare del prestito o della linea di credito; condizioni peggiorative vengono poi applicate anche sulle scadenze e sulle garanzie richieste dalle banche.

In particolare, appare necessario accrescere fortemente la capacità del sistema bancario di valutare il *rating* tecnologico delle imprese, il contenuto innovativo dei progetti e i relativi potenziali ritorni sull'economia.

ancora una volta - come è stato già evidenziato - ci troviamo nella situazione paradossale di una discussione avulsa da un provvedimento per il quale è stata posta la questione di fiducia, negando nuovamente le prerogative proprie del Parlamento e con esse gli spazi

Mi riferisco, in particolar modo, alle norme introdotte all'articolo 7, riguardanti in maniera significativa il settore dei trasporti e delle infrastrutture. Il comma 3-*bis* dell'articolo 7, inserito durante l'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, introduce alcune modifiche all'articolo 20 del decreto‑legge 185 del 2008, proprio recentemente convertito in legge, in materia di norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale. In particolare, la lettera *a)* attribuisce al commissario i poteri sostitutivi degli organi ordinari e straordinari; a tal fine, egli può derogare ad ogni disposizione vigente, nel solo rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento dei contratti contratti pubblici nonché dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico. In sostanza, la disposizione ricalca la norma relativa al cosiddetto super commissario del modello protezione civile, cui sono attribuiti i poteri connessi allo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, ed estesi, ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 343 del 2001, ai grandi eventi. Tali poteri consentono ai commissari di agire per mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, con il solo limite del rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Insomma, con la nuova procedura viene meno il vincolo esplicito al rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, nonché di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale. La norma, come si comprende agilmente, tende a trasformare l'ordinario in straordinario e, di conseguenza, l'efficienza, che da tempo - verrebbe da dire, ovunque nel nostro Paese - non costituisce più una prassi, diventa esclusiva prerogativa di emergenza e poteri eccezionali. È una cultura dell'emergenza - e viene da dire - dello Stato militare, di polizia, che progressivamente state sostituendo ad uno Stato che state invece smantellando inopinatamente, senza far applicare le leggi che ci sono e, di conseguenza, farle rispettare. Così pure il comma 3-*ter* dell'articolo 7 che prevede che i contratti di servizio relativi al trasporto pubblico ferroviario abbiano una durata minima non inferiore ai sei anni, rinnovabili di altri sei;

proprio perché l'8a Commissione del Senato - il presidente Grillo è qui presente - stava conducendo un pregevole lavoro di audizioni con i vertici di Ferrovie e con le Regioni, finalizzato proprio ad un atto di indirizzo in tal senso, ma di certo più organico e, soprattutto, direi più rispettoso e, forse, mi permetto, anche più persuasivo nei confronti delle Regioni che, lo ricordo, hanno in tale materia poteri concorrenti a quelli dello Stato.

che sono davvero ingiustificate e ingiustificabili. Infine, all'articolo 7-*octies* si riconosce l'opportunità di una somma modesta e, peraltro anche discutibile, al risarcimento, neppure simbolico, nei confronti degli obbligazionisti di Alitalia; un risarcimento che prevede ancora una volta la copertura del fondo previsto con l'impiego improprio e sciagurato dei fondi FAS per le aree sottosviluppate. Ci sarebbero stati, invece, margini per modificare le fonti di copertura e dare maggior consistenza e differente natura a quei dovuti risarcimenti; magari sostituendo - come avremmo proposto - le vecchie obbligazioni con le nuove emissioni dei titoli di Stato e impiegando nei termini più congrui e previsti i fondi FAS. La vicenda Alitalia, colleghi, non è chiusa e meno che mai si chiude con questo atto. Ritorneremo, alla ripresa della pausa pasquale, sul tema che riguarda i lavoratori di Alitalia, quelli in cassa integrazione che non hanno ancora ricevuto l'indennizzo dovuto nonostante i mesi passati; quelli che, nonostante le tutele al reddito, rischiano comunque la perdita di abilitazione al volo; quelli che, per incapacità sostanziale dell'improvvisato *management*, rischiano il licenziamento dalla nuova compagine, che per quanto alleggerita e ridotta continua inesorabilmente a perdere quote significative di mercato e con esse entrate necessarie per l'equilibrio di bilancio, davvero ancora molto lontano.

Commissioni competenti erano impegnate con il lavoro proprio e ordinario, i cui intuibili esiti lasciavano prefigurare una possibile convergenza degli obiettivi e di certo una più organica e precisa definizione della norma, ma anche un maggior rispetto dei rapporti istituzionali.

Evidentemente, così non è avvertito da questo Governo, che utilizza il Parlamento come un proprio scendiletto e che può disporre - e lo fa - di una maggioranza plaudente e al suo servizio, pronta a ricevere acriticamente quanto il *dominus* chiede ed ordina. L'alterazione sistematica e lo stravolgimento costante delle prassi e delle procedure istituzionali rendono il Parlamento nei fatti - ancor prima che nel giudizio - anziché una risorsa a disposizione del Paese, un intralcio un ingombro da evitare finché possibile, o da saltare quando l'impatto è reso inevitabile dalle norme ancora vigenti. Così facendo e continuando, il giudizio di inutilità, di spreco delle risorse pubbliche*,* nonostante i nostri rutilanti affanni, sarà a breve - se già non lo è - inesorabile nell'opinione pubblica e nel giudizio prevalente del Paese.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, siamo ormai al sesto provvedimento sulla crisi: ancora una volta, ci troviamo di fronte un provvedimento insufficiente a fronteggiare una crisi economica e sociale che rischia di essere devastante

reale opportunità di ripresa. Tanta fretta da porre addirittura la questione di fiducia, mentre è ancora in discussione il disegno di legge n. 1195, che, tra l'altro, contiene alcune norme che si sovrappongono o rischiano di sovrapporsi a quelle inserite in questo decreto-legge: penso al tema dei distretti industriali e delle reti d'impresa. Molto di più si sarebbe potuto fare, ad esempio, sul terreno degli ammortizzatori sociali e del sostegno al reddito: per quanto riguarda gli anziani e le fasce deboli della popolazione, più che le facilitazioni per il *decoder* sarebbero stati utili interventi di contrasto alla povertà, di sostegno al reddito e soprattutto di salvaguardia dei servizi sociali essenziali. Per quanto riguarda le prestazioni occasionali di tipo accessorio, questa poteva essere un'occasione per fare chiarezza, facendo emergere una parte di lavoro nero e dando una possibilità vera ai giovani di cominciare a entrare nel mondo del lavoro, anche utilizzando la rete del volontariato italiano le organizzazioni sociali e culturali: anche questa norma, però, è insufficiente, confusa ed estremamente limitata. Pur avendo apprezzato quella parte del decreto-legge che propone misure di semplificazione delle procedure relative agli ammortizzatori sociali, l'aumento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, gli incentivi per l'auto e per i veicoli non inquinanti gli aiuti ai settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, dobbiamo purtroppo constatare che le risorse messe a disposizione sono ancora una volta troppo poche spesso ripagate dalle stesse imprese in termini di maggiori entrate da loro recuperate e riduzioni di spese relative a investimenti a loro favore. negativo anche il fatto che si continui ad attingere ai fondi FAS, sottraendo ingenti risorse finanziarie per lo sviluppo del Mezzogiorno. Questa disattenzione per le sofferenze delle persone, per le difficoltà delle piccole e medie imprese e per le aree deboli del nostro Paese fa sì che il giudizio sul decreto-legge anticrisi non possa che essere negativo. Dopo mesi di ottimismo, il Presidente del Consiglio ha quasi ammesso nei giorni scorsi che anche l'Italia è in crisi. Fino a qualche giorno fa eravamo l'unico Paese baciato dalla fortuna: noi non avevamo problemi. Tuttavia l'economia italiana è entrata in recessione già dal secondo trimestre del 2008. Da allora, abbiamo registrato un vistosissimo calo della produzione industriale, la chiusura di molte aziende, l'aumento del ricorso alla cassa integrazione, il calo delle esportazioni, la crescita della disoccupazione; interi settori sono entrati in grave difficoltà. L'insieme di questi fattori ha avuto ripercussioni negative sulla distribuzione dei redditi, sulle buste paga; basti pensare alla perdita di posti di lavoro, all'ulteriore restrizione delle possibilità occupazionali dei giovani. I poveri si sono ulteriormente impoveriti. Consapevoli di ciò, abbiamo presentato proposte tese a sostenere i settori più deboli della società italiana e le piccole e medie imprese. In modo particolare abbiamo cercato di porre all'attenzione del Governo la grave situazione di crisi del settore del turismo, uno dei settori ancora trainanti della nostra economia, peraltro così sottovalutato dalla maggioranza. Fra un mese circa comincia la stagione turistica estiva. I dati del 2008 e i primi dati del 2009 fanno impressione. La perdita è secca e si va ad aggiungere al continuo scivolamento verso il basso della nostra economia turistica, che dura ormai da qualche anno. In questi anni di crisi si è aperto un contenzioso tra Stato, Regioni e concessionari demaniali, i quali hanno proposto di rivedere la normativa vigente in materia di canoni concessori, ritenuti troppo pesanti vista la restrizione dei mercati turistici. Gli operatori balneari pongono con forza il problema di rivedere complessivamente una disciplina che punisce chi più investe e favorisce chi ha posizioni di maggior favore nell'ambito delle concessioni demaniali, parificando un po' tutto verso l'alto. Le richieste dei concessionari erano confluite in un accordo tra il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al turismo,

che promettere iniziative mirabolanti anche nel settore del turismo, per distogliere in realtà l'attenzione dal fatto che intanto, con la manovra di bilancio, si tagliavano pesantemente le già esigue risorse destinate al turismo stesso. Non solo, i 48 milioni che il Governo Prodi aveva destinato al settore sono stati distolti dalle loro finalità originarie concordate con le Regioni, ovvero l'innovazione del settore turistico-alberghiero, per finanziare non meglio precisati progetti di eccellenza. Si tagliano i soldi all'ENIT e nello stesso tempo, con la scusa di ridurre il numero di consiglieri di amministrazione, si punta in realtà al commissariamento dell'Agenzia nazionale per il turismo. Infine, di fronte al nostro emendamento teso a risolvere l'eterno contenzioso tra demanio e concessionari demaniali e a prevedere misure dei canoni di concessione più contenute, una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, in modo da calmierare i prezzi e facilitare l'aumento dell'afflusso di turisti, si è risposto ancora una volta no: parere contrario del relatore, Governo conforme. Abbiamo inoltre proposto di introdurre un credito d'imposta finalizzato alla rottamazione degli arredi, della biancheria, dei tessuti degli alberghi e delle altre strutture ricettive per consentirne la riqualificazione, e un emendamento teso ad armonizzare le aliquote IVA applicate alle imprese turistiche al 7 per cento, avvicinandole a quelle europee visto che quelle italiane sono tra le più alte. Ma, anche in questo caso: parere contrario del relatore, Governo conforme. Questo ripetuto ritornello è lo specchio del tipo di collaborazione che la maggioranza ci offre. Davvero si pensa che un settore come il turismo, che potrebbe essere rilanciato e costituire un'ancora di salvezza per la nostra economia e per l'occupazione, possa rimanere fuori da un decreto-legge che affronta proprio il problema dei settori in crisi? E in generale essere escluso da tutti i provvedimenti finora adottati? Che senso ha allora pensare al ripristino di un Ministero del turismo e fare accordi-quadro che non trovano mai una effettiva applicazione? Ancora *spot*, enunciazioni ad effetto, ma ben poco di concreto: tanti protocolli d'intesa inesorabilmente disattesi.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, nell'affrontare la discussione sulla fiducia al disegno di legge di conversione del decreto-legge oggi in esame sono tante le motivazioni che mi spingono ad esternare quel senso di disagio e di delusione che da alcuni mesi sta diventando sempre più acuto e profondo. Innanzitutto, i tempi. In una esigua manciata di ore in questa Aula - e in pochi minuti in Commissione - ci troviamo costretti a discutere ed approvare un testo che contiene interventi che coprono le tre aree più sensibili agli effetti negativi della crisi in atto: imprese, lavoratori (quindi famiglie) ed enti locali. È esattamente il contrario della serietà che il nostro ruolo imporrebbe e che il momento drammatico esigerebbe. In secondo luogo, le regole istituzionali per l'ennesima volta calpestate e sfregiate. È impressionante osservare il cammino dei decreti-legge che il Governo ha emanato in questi mesi. Preceduti da annunci roboanti, che di volta in volta creano nel Paese aspettative fuori misura, i testi, strada facendo, raccolgono di tutto, per diventare infine una sorta di contenitore *omnibus*, mancando così di organicità e di chiarezza rispetto agli obiettivi che ci si pone. Stavolta però credo si sia superato il limite, con l'assorbimento nel decreto in esame di un altro decreto-legge, quello sulle quote-latte, che si stava avviando verso la non conversione in legge, grazie alla convinta battaglia delle opposizioni, delle associazioni di categoria e delle migliaia di allevatori e agricoltori che chiedevano a gran voce un ripensamento nel segno della legalità, dell'equità e del rispetto delle regole. Ci eravamo illusi che potesse esserci un sussulto di buon senso, che potessero prevalere l'ascolto e il confronto, in modo da risolvere la questione senza alimentare ulteriori tensioni e senza umiliare chi si è mosso dentro la legge. Invece no. Avete scelto la strada della forzatura, assegnando la questione delle quote-latte ad un provvedimento estraneo al settore agricolo, uscendo da ogni logica e prassi parlamentare, il tutto condizionato dalla necessità di chiudere contrasti ed esigenze divergenti in seno alla maggioranza stessa. Nel merito, restano pertanto valide per noi tutte le argomentazioni e le critiche espresse in sede di approvazione qui al Senato di quel decreto-legge, oggi diventato maxiemendamento all'interno di qualcos'altro. Tempi e regole, quindi, ma soprattutto il motivo vero del disagio cui accennavo è il fatto che l'oggetto di questo decreto-legge è la crisi e lo è per la sesta volta in pochi mesi; è il fatto che le risposte vengono date, come tutte le altre volte, in maniera frammentata, parziale, disorganica, tardiva - quello sugli incentivi alle auto ne è un esempio - quindi inefficace, inadatta e insoddisfacente. È l'assenza di risposte al dramma di migliaia di lavoratori che vedono ridotto il proprio reddito se non addirittura la mancanza di lavoro. Oggi i giornali ci parlano dei dati sul ricorso alla cassa integrazione ordinaria, cresciuta a marzo del 925 per cento rispetto ad un anno fa;

Tutti sappiamo bene che, oltre a questi dati, vi sono migliaia di persone che non ricadono in queste statistiche e sono coloro per i quali il diritto alla tutela del reddito non è previsto. In questa situazione faccio un appello: la si smetta di fare propaganda e annunci cui non seguono atti concreti rispetto ad un problema estremamente serio, rispetto a chi oggi sta pagando il prezzo più alto della crisi. È inaccettabile che in questi mesi si sia continuamente parlato in televisione e sui giornali di 9 miliardi di euro a sostegno del reddito, di estensione degli ammortizzatori sociali a chi non ha tutele previste dall'ordinamento, quando in realtà quei lavoratori non riscuotono un euro da qualche mese. Cosa diciamo loro? Continuiamo a dire di aspettare? E intanto le norme sono sempre più confuse, pasticciate, si sovrappongono le une alle altre in maniera incoerente e incomprensibile. Si è tuttora in attesa dei provvedimenti attuativi, proprio nel momento in cui la crisi sembra stia raggiungendo il suo picco più alto. Da qui la proposta del Partito Democratico di misure immediate, secche, chiare, inclusive

nessuno. A questo s'intreccia la questione relativa agli enti locali. Ne ha parlato molto bene il senatore D'Ubaldo e quindi non mi soffermo sul significato di tutto il suo intervento, teso ad evidenziare come la rinegoziazione del Patto di stabilità interno possa essere veramente una leva per gli investimenti e uno strumento di rilancio per l'economia. Voglio soffermarmi su un'altra questione. Oggi i Comuni sono in prima linea a dover far fronte all'onda d'urto dell'impoverimento incipiente di migliaia e migliaia di cittadini. È del tutto evidente che nei Comuni si sta verificando una sorta di imbuto della domanda sociale. È del tutto evidente che le famiglie che vanno in difficoltà si stanno rivolgendo ai Comuni chiedendo aiuto e sostegno e che questa domanda richiede interventi solleciti, forti e incisivi da parte delle amministrazioni pubbliche. Tanti sono i Comuni che, nonostante le gravi difficoltà economiche, hanno approvato e stanno approvando piani e pacchetti anticrisi. Ma fino a quando reggeranno? Fino a quando potranno sopportare interventi che, da una parte, stanno mettendo a dura prova la loro autonomia finanziaria e, dall'altra, hanno operato tagli pesanti sui fondi per le politiche sociali e, aggiungo, sulle politiche per la scuola, veri strumenti e opportunità per uscire dalla crisi? Quale politica anticrisi è questa? Si pensa forse che un taglio degli organici di 4.000 posti in Lombardia non ricadrà sulle politiche che gli enti locali dovranno mettere in campo nel prossimo anno scolastico? Il malessere sta crescendo. Un movimento di protesta trasversale sta caratterizzando l'azione di tanti sindaci che si sentono traditi. Un giorno si approva all'unanimità una mozione sulla rinegoziazione del Patto di stabilità interno, il giorno dopo s'inserisce un emendamento che invece è ben lontano dalle necessità reali del Paese. Signor Presidente, come Partito Democratico abbiamo fatto proposte serie, fattibili, concrete. avremmo potuto affrontare anche la discussione su questo provvedimento con approfondimenti che credo sarebbero stati interessanti, ma, ancora una volta, ci è stato impedito dalla richiesta di fiducia da parte del Governo; ancora una volta, le nostre proposte vengono scartate *a priori*. Continueremo comunque con la nostra azione di opposizione determinata e responsabile che ha a cuore gli interessi generali del Paese. Signor Presidente, gentili colleghi senatori, onorevole Sottosegretario, questo provvedimento ha come obiettivo quello di introdurre delle misure urgenti a favore dei settori industriali in crisi. La strada intrapresa fino ad oggi ha portato all'adozione di un pacchetto di aiuti che in prima analisi sembra avere un raggio di intervento abbastanza limitato, concentrandosi in primo luogo a risollevare le sorti delle imprese che operano nel settore dell'automobile, attraverso la concessione di incentivi per il rinnovo del parco circolante. Questo non significa assolutamente che esistono settori di serie A o di serie B, ma semplicemente che il comparto dell'automobile è forse quello che coinvolge un maggiore indotto. Ulteriori risorse andranno infatti alle imprese dei distretti del settore tessile, moda e calzature, settori che hanno sempre fatto del nostro Paese un punto di riferimento in tutto il mondo. Grazie ad un lavoro svolto in Consiglio dei ministri e poi, durante possiamo parlare anche di tutti questi settori che rimarcano e testimoniano la qualità dei nostri prodotti. L'articolo 2 consente, per esempio, una detrazione del 20 per cento delle spese sostenute da febbraio a dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, energetica, nonché apparecchi televisivi e computer, in favore dei contribuenti che fruiscono della detrazione IRPEF del 36 per cento per interventi di ristrutturazione edilizia effettuati a partire dal 1° luglio 2008. Oltre alla conferma e all'ampliamento delle misure incentivanti, sono state poi inserite norme molto importanti per il sistema delle imprese. In particolare, si introduce la regolamentazione delle reti d'impresa con rilevanti benefici in tema di capacità innovativa e competitività sul mercato. Un'altra misura importante è l'avvio concreto del Fondo di garanzia per le piccole medie imprese, che rappresentano la spina dorsale del nostro sistema economico; un Fondo di garanzia che può disporre complessivamente di 1,6 miliardi di euro.

Aiuteremo quindi esclusivamente quelle imprese che decidono di rimanere sul nostro territorio impegnandosi così a sostenere l'economia del Paese anche nei momenti di crisi. Ricordiamo poi il dibattito in materia di Patto di stabilità, in merito al quale anche in questi casi è stata la Lega Nord a chiedere che per i Comuni virtuosi vi fossero delle possibilità in più per spese di investimento per la sicurezza e per il pagamento dei fornitori.

e la possibilità che il Ministero disponga del pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento straordinario di integrazione salariale, quando per l'impresa ricorrano comprovate difficoltà di ordine finanziario accertate dall'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente. In questo caso, con la previsione che tale pagamento dovrà avvenire contestualmente all'autorizzazione al trattamento, nonché con la previsione - in via sperimentale per il periodo 2009/2010 - del pagamento anticipato da parte dell'INPS anche per la cassa in deroga. Non solo: il provvedimento pone dei requisiti ai fini dell'accesso alla cassa integrazione in deroga ed alla mobilità in deroga, disponendo che l'ammissione del lavoratore è subordinata al conseguimento di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 90 giorni ovvero, nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale, un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi. Il lavoro deve però essere incentivato anche attraverso, per esempio, l'assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga.

La crisi finanziaria che sta interessando questo periodo epocale è solo una parte di una crisi più complessa che vede le sue origini non solo nel crollo dell'economia statunitense, ma anche nella parola globalizzazione.

è stata sicuramente lanciata troppo presto, nel senso che non eravamo pronti, né avevamo gli strumenti per affrontarla, tutti fattori che ci hanno esposto ad un debito troppo elevato. L'attuale legislatura, che ci vede qui da quasi un anno, è iniziata con una pesante responsabilità: l'impegno assunto per l'applicazione del Patto di stabilità, quello che, per intenderci, ha prodotto i ritardi dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione nei confronti di aziende private, però la cifra era stata calcolata modificando solo i tendenziali di PIL e quelli del deficit, che non tendeva allo zero, Inutile poi negare la forte preoccupazione generata da una pluralità di fattori che hanno inciso negativamente sul mercato. Tra questi sicuramente la mancanza di trasparenza dei bilanci delle banche, le valutazioni non tempestive delle agenzie di *rating* sul deterioramento delle condizioni economiche degli intermediari. A questi si aggiunge la violazione di regole prudenziali da parte delle banche nell'utilizzo di strumenti finanziari derivati. Nel settore finanziario globale, rispetto al tradizionale assetto basato sull'attività delle banche, è aumentato enormemente il peso dei mercati e degli intermediari non bancari e questo costituisce un elemento fondamentale per spiegare alcuni aspetti della crisi.

ore a disposizione per discutere di tutto ciò. La stessa maggioranza che sostiene il Governo ritiene inutile e non dignitoso intervenire in questo dibattito. Siamo di fronte all'ennesimo decreto-legge che costringe i tempi della discussione parlamentare che viene suggellata dall'ennesimo voto di fiducia.

un decreto-legge o almeno parti di esso decadute. Siamo davvero di fronte ad un paradosso istituzionale che credo crei un grave *vulnus* nell'autonomia del Parlamento. insomma, all'ennesimo contributo che questo Governo, supinamente sostenuto dalla sua maggioranza, sta dando ad un progressivo spostamento di quello che è uno dei poteri sanciti dalla Costituzione, quello legislativo, che viene vieppiù assorbito dal potere esecutivo. Su questo dovrebbero levarsi non solo le grida dell'opposizione, ma anche una riflessione attenta delle forze più responsabili del Governo, delle istituzioni, della stessa maggioranza. Se questo processo va avanti con tale velocità, così come sta accadendo in questi mesi, credo che davvero siamo di fronte ad una Costituzione che viene nei fatti mutata, determinando gravi ripercussioni sull'autonomia dei poteri in essa sanciti.

a noi, all'opposizione, di intervenire nel merito con un confronto sull'articolato del decreto-legge in esame. Signor rappresentante del Governo, ci viene impedito finanche di apprezzare quelle parti del provvedimento che abbiamo sostenuto nella discussione parlamentare nell'altro ramo del Parlamento, alla Camera, e che abbiamo contribuito a migliorare. Avremmo voluto andare anche oltre nella discussione svolta nelle Commissioni competenti e anche nella stessa Aula del Senato, se questo ci fosse stato consentito. Ma così non è Vorrei ricordare, entrando nel merito, che siamo di fronte ad un provvedimento che riguarda la crisi più grave che il nostro Paese sta vivendo da molti decenni a questa parte. Eppure è una crisi che viene da lontano. La recessione in cui l'economia italiana è entrata non data oggi, non data qualche mese, ma data ormai più di un anno. Era il secondo trimestre del 2008 quando i primi dati indicavano che il sistema economico del nostro Paese si avviava verso una grave recessione.

abbiamo visto calare quello che negli anni passati era stato uno dei livelli di eccellenza della nostra economia, le esportazioni. Infine, cresce, arrivando pericolosamente alla doppia cifra, la percentuale di disoccupati nel nostro Paese ed intere filiere produttive sono entrate in un vorticoso giro di difficoltà.

che da anni viene denunciata dai maggiori centri di osservazione - continua ad aumentare e che cresce la percentuale delle famiglie sotto la soglia di povertà. Non si tratta di creare allarmismi, ma di prendere atto del quadro vero dell'economia reale, della vita quotidiana di tante famiglie, di tante imprese e di tanta parte del nostro Paese. Avere consapevolezza di ciò significa avvertirne la responsabilità e avere chiare le priorità nell'azione di Governo.

Parimenti, l'altro filone di intervento avrebbe dovuto essere rappresentato dal sostenere le condizioni per la fuoriuscita dalla crisi. Il tempo non è una variabile indipendente,

c'è bisogno di provvedimenti veloci, chiari e seri, nonché di risorse adeguate. Voglio ricordare come l'Italia abbia messo a disposizione, mettendo insieme i vari decreti e

che altri Paesi, con economie non dissimili dalla nostra, hanno voluto mettere in campo con una consapevolezza che il nostro Governo ha inteso non manifestare. C'è stata una sottovalutazione voluta e, vorrei dire, vorrei dire, quasi ideologica e schizofrenica. Ho sentito spesso in questi mesi richiamare il merito del ministro Tremonti; noi lo abbiamo riconosciuto abbiamo riconosciuto quando alcuni mesi fa ebbe a denunciare il rischio di questa crisi che si sarebbe riverberata nell'economia del nostro Paese. Quel merito però è rimasto lì,

di cosa ha potuto godere in questi mesi da questi provvedimenti? Una piccola e media impresa, che ha visto chiudersi le sue linee di credito o ostacolare la sua possibilità di crescere sui mercati internazionali o ridursi fortemente il suo mercato interno, di quale provvedimenti ha potuto godere concretamente in questi mesi? Se ci facciamo queste domande e rispondiamo onestamente, abbiamo il segno di come i pur numerosi provvedimenti che il Governo ha adottato hanno mancato di coraggio, di concretezza e di consapevolezza della gravità della crisi che il nostro Paese ha davanti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per porre all'attenzione di questa Assemblea un fatto che giudico di estrema gravità per le implicazioni politiche connesse. Mi riferisco all'atto di orientamento con cui il Ministero dell'interno, per il tramite della prefettura di Perugia, ha invitato il Comune della stessa città a riformare i propri statuti e regolamenti in materia di circoscrizioni di decentramento entro la data di convocazione dei comizi elettorali del prossimo 23 aprile, il tutto con espressa indicazione che in caso contrario, qualora il Comune di Perugia non intervenga in tal senso, il Ministero ritiene che debbano essere indette le elezioni soltanto per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Queste dichiarazioni sono state esternate al Comune di Perugia con una lettera inviata dal prefetto al presidente del consiglio comunale il 2 aprile scorso. È grave, onorevoli colleghi, che con questo atto il Ministero intervenga con una tempistica che, evidentemente, impedisce al Comune di Perugia di modificare il proprio statuto nei termini indicati, è ancora più grave il fatto che il Governo, attraverso questo atto, anticipi l'intenzione di emanare un provvedimento che andrebbe a ledere l'autonomia del Comune e del consiglio comunale, intervenendo su un legittimo atto amministrativo di riforma delle circoscrizioni adottato dal Comune di Perugia in attuazione della legge approvata nella scorsa legislatura, portando il numero delle circoscrizione da 13 a 5. Evidenzio, inoltre, che con un provvedimento del genere il Governo impedirebbe ai cittadini di avvalersi liberamente del sacrosanto diritto di partecipare alle elezioni in maniera democratica. A ciò si aggiunga che le motivazioni addotte nell'atto di orientamento, oltre a non essere fondate, vanno ad inficiare il principio di autonomia dei Comuni nel determinare i propri assetti statutari e, comunque, dovrebbero eventualmente essere avanzate all'interno di un atto che avvia un procedimento giurisdizionale, essendo l'autorità giudiziaria l'unica legittimata a decidere sulle argomentazioni che sono alla base dell'orientamento del Ministero. In conclusione, colleghi, si tratta di una impropria e illegittima ingerenza istituzionale che non ha precedenti nella storia della nostra democrazia ed io, insieme ai miei colleghi dell'Umbria del Partito Democratico - è qui presente il senatore Agostini chiedo ed auspico che il Governo e, in particolare, il Ministro dell'interno al quale abbiamo chiesto un incontro urgente a tale proposito, muti l'orientamento espresso o, comunque, non vi dia seguito al momento della convocazione dei comizi elettorali.